Ministro della transizione ecologica sui recenti ulteriori rincari del costo dell'energia e sulle misure del Governo per contrastarne gli effetti». Ricordo che è in corso la diretta televisiva con la RAI.

il secondo è un'analisi, anche se abbastanza rapida, delle misure per incrementare la sicurezza del sistema nel breve e medio termine;

si è ridotta sostanzialmente, in parte a causa del calo naturale dei giacimenti e del fatto che non si sono effettuati nuovi investimenti in ricerca e produzione. I numeri parlano numeri parlano di poco più di 15 miliardi di metri cubi prodotti nel 2001 contro i 3 miliardi di metri cubi prodotti oggi. Questo vuol dire che si è passati

Nel nostro *energy mix* sostanzialmente abbiamo gas e rinnovabili, quindi questo sancisce una fortissima dipendenza dall'importazione. Le importazioni dalla Russia, per il caso di specie attuale, sono incrementate in valore assoluto e in percentuale da 20 miliardi di metri cubi - il 25 per cento dei consumi - nel 2011 a 29 miliardi di metri cubi nel 2021, che equivale a circa il 38 per cento dei consumi. Questa è la nostra attuale dipendenza dalla Russia. Dal punto di vista delle infrastrutture di importazione, abbiamo un sistema di approvvigionamento e di trasporto diversificato che è abbastanza resiliente, soprattutto rispetto agli altri Stati membri, ed è alimentato prevalentemente con gas prodotto all'estero, come dicevo poc'anzi,

connettendosi alla rete nazionale dei gasdotti a Tarvisio. Qui passano i 29 miliardi di metri cubi dell'ultimo periodo che provengono dalla Russia, circa il 40 per cento del nostro *import.*

Il gasdotto permette l'importazione - e addirittura, in alcuni giorni prima della crisi, un po' di esportazione di gas dall'Italia - del gas proveniente dal mercato nordeuropeo, un *mix* di gas che proviene da Norvegia, Olanda, Danimarca e Regno Unito e anche di gas naturale liquido importato attraverso terminali di rigassificazione nordeuropei.

attualmente trasporta il 3 per cento del nostro gas (2,2 miliardi di metri cubi). Potrebbe portarne 12 miliardi, ma il punto è che non riceviamo molte forniture dal Nord Europa, che soprattutto in un momento come questo tende a internalizzare sul proprio

è grosso: sono oltre 21 miliardi di metri cubi e potrebbe arrivare a 27 miliardi, pertanto ha ancora un po' di capacità sfruttabile. Il gasdotto Greenstream connette la rete nazionale dei gasdotti a Gela e importa nel nostro Paese il gas prodotto in Libia: questo è massimizzato, perché va direttamente ai punti di produzione, e trasporta 3,2 miliardi di metri cubi (circa il 4 per cento). Infine, Adriatic pipeline (TAP), che interconnette Italia, Grecia e Albania, come sapete, e si connette alla rete nazionale dei gasdotti a Melendugno, in Puglia, trasportando - tramite la Turchia - il gas che proviene dall'Azerbaijan. Questa è l'ultima infrastruttura di *import* realizzata, come ricorderete tutti, entrata in funzione nel novembre 2020; trasporta attualmente il 10 per cento del nostro gas, pari a circa 7 miliardi di metri cubi, e potrebbe arrivare all'incirca a 8,5 con l'attuale assetto. Ci sono poi tre rigassificatori: uno a Panigaglia (l'unico in terraferma) e due *off-shore* installati al largo nella zona di Rovigo e nella zona di Livorno. Questi producono il 13 per cento del nostro gas per circa

Di questo sistema - composto quindi da tre stazioni di rigassificazione e cinque gasdotti - fa parte qualificante anche la serie di giacimenti di stoccaggio di gas naturale. Ricordo che, per assicurare il bilanciamento di consumi tra inverno ed estate - non è quindi solo un problema di valore medio: ci sono periodi di picco e altri, come l'estate, in cui il bisogno è inferiore cui il bisogno è inferiore - disponiamo di 18 miliardi di metri cubi, una parte dei quali è destinata allo stoccaggio strategico, producibile solo in caso di emergenza prolungata, e circa 12 miliardi di metri cubi sono destinati allo stoccaggio commerciale di gas di proprietà dei *trader*. La parte che rimane è, appunto, una riserva strategica proprietà delle imprese di stoccaggio e può essere erogata in condizioni di emergenza prolungata, a tutela residuale del settore civile. civile. Con questo assetto - credo che i numeri siano abbastanza chiari - vediamo gli scenari di possibile interruzione delle forniture di gas dalla Russia, nell'ipotesi in cui a un certo momento si chiuda il rubinetto. È importante sottolineare che in questo momento il flusso di fornitura attraverso la Russia è il più alto registrato in tempi recenti. La fornitura è assolutamente costante in tutta Europa; anzi, si è sollevata - come penso abbiate sentito - una riflessione sul fatto che comunque l'Europa sta continuando ad acquistare il gas e la fornitura in questo momento è continua, e questo porta a pagamenti di un ordine di grandezza di circa un miliardo di euro al giorno di acquisto da parte dell'Europa. In un momento, purtroppo, di guerra come questo, capite che la cosa ha implicazioni che vanno oltre il settore energetico: noi (Europa)

Supponiamo che possa esserci un'interruzione: nel breve termine, cioè fra un mese, come ordine di grandezza, grazie all'atteso miglioramento delle condizioni climatiche, si stima una riduzione della domanda per uso civile dell'ordine di 40 milioni di metri cubi al giorno. Questo è quello che succede quando il tempo migliora, come in questo periodo (fine marzo), assumendo che ci siano condizioni di freddo *standard*, quindi non un picco invernale ritardato. Pertanto, anche una completa interruzione dei flussi dalla Russia da questa settimana non dovrebbe comportare problemi di fornitura interna. Eventuali picchi di domanda potrebbero essere assorbiti modulando opportunamente i volumi di stoccaggio residui - il nostro attuale residuo è circa il 25 per cento di quello che avevamo a inizio inverno, un po' meno del solito in questa stagione, ma siamo tutti partiti in Europa con meno stoccaggio Europa con meno stoccaggio - e con le altre capacità di importazione non dovremmo avere alcun tipo di problema. Problemi per assicurare la fornitura a tutti i consumatori italiani in questo scenario potrebbero avvenire solo in caso di un picco di freddo eccezionale a fine marzo o un contestuale evento catastrofico (*disruptive*) su altre rotte di importazione, che in questo momento non abbiamo motivo nemmeno di considerare. Vediamo il medio termine, che è oggettivamente la parte più preoccupante.

L'attivazione - si spera con successo - delle misure di breve e medio termine descritte nel seguito, e che fra poco vi illustrerò, anche con alcune norme che sono in corso di pubblicazione, dovrebbe mitigare la criticità che oggi è essenzialmente legata al prezzo. Qui vengo alla nota dolente. In questo momento, a marzo del 2022, ci siamo attestati a un prezzo medio di 1,50 euro per metro cubo. Quindi, per essere molto chiaro, se dovessi stoccare 10 miliardi di metri cubi, mi servirebbero 15 miliardi di euro. Sto facendo un calcolo un po' vuoto per pieno, ma credo sia evidente. Quindi, chi fa questo stoccaggio deve mettere 15 miliardi sul tavolo. Vi faccio presente che un anno fa, di questi tempi, quando il gas era esattamente uguale a quello che c'è adesso, anzi un po' di meno, perché ora stanno flussando leggermente di più, il costo era di 30 centesimi a metro cubo. Quindi, gli stessi 10 miliardi avrebbero richiesto un anticipo di 3 miliardi. Ora, non ho nessuna intenzione di sollevare problemi senza proporre soluzioni, come qualcuno ha voluto intendere; però, siccome la quantità di gas è uguale, non è molto giustificato non è molto giustificato il fatto che, a parità di tutto, il prezzo mi vada da 30 centesimi a 1,5 euro e quindi che uno stoccaggio mi costi da 3 miliardi di anticipo, che potrà fare l'operatore, a 15 miliardi, perché è una cosa un po' diversa. Questa è stata la mia affermazione, forse un po' dura e sicuramente non mi sono espresso con termini giuridicamente corretti, ma credo abbiate capito lo spirito: se la materia è la stessa, non è possibile costi cinque volte di più, perché stiamo mettendo in ginocchio gli operatori, i cittadini e tutti quanti. È ovvio che non c'è qualcuno che in Italia sta facendo una cosa sbagliata. È un problema di quotazione di un mercato di questi *hub,*

stiamo monitorando con la Commissione europea ogni aspetto e abbiamo tutti i grafici dell'evoluzione del prezzo del gas e, ovviamente, dell'elettricità. Come sapete, infatti, e lo vedremo fra un attimo, il gas con il marginale determina il prezzo dell'elettricità. C'è questa crescita continua e poi si vede che, il giorno in cui scoppia il conflitto, i grafici hanno un'impennata. un'impennata. Sulla stampa internazionale sono state fatte anche osservazioni sul fatto che ci possano essere influenze su queste quotazioni da parte addirittura dei produttori russi. Questi sono argomenti molto delicati a livello internazionale. Li stiamo trattando in Commissione e abbiamo parlato con il gabinetto della presidente Von Der Leyen già due volte e vi illustrerò alcune proposte operative. Certo è che, senza bisogno di essere un giurista o un esperto, oggi

tanto. Il problema sul medio termine, dunque, è lo stoccaggio. Stiamo operando e vi descriverò dopo alcune misure che stiamo cercando di portare avanti per mitigare e accelerare gli stoccaggi. Nel lungo termine, quindi dal prossimo inverno in poi,

ampliarla. Chiaramente un triennio è il periodo minimo per avere un inizio di diversificazione completa,

Come dicevo poc'anzi, il mercato del gas naturale al punto di scambio virtuale (PSV) in Italia, a seguito dei numeri di cui vi parlavo prima, è passato da 20 euro al megawattora, che corrispondeva a 20 centesimi al metro cubo, nel gennaio del 2021, fino a circa 160 euro al megawattora, che è corrisposto a 1,7 euro per metro cubo. Ricordatevi il calcolo degli stoccaggi e quindi vedete la relazione tra il problema sullo stoccaggio e quello sulle bollette e, per ovvi motivi, sulle attività industriali.

Per quanto riguarda i prezzi dell'energia elettrica all'ingrosso, il prezzo unico nazionale (PUN) ha registrato valori *record*. Nelle ultime settimane si sono raggiunti i valori più elevati da quando la Borsa italiana è stata costituita: si sono superati i 600 euro al megawattora. Negli ultimi giorni i valori si sono attestati intorno a 300 euro al megawattora, anche come diretta conseguenza dei prezzi del gas naturale, che determinano il costo marginale degli impianti di generazione elettrica a gas. Per essere chiari, per essere del tutto indipendenti dal gas,

Non si tratta di un fenomeno italiano, ma di andamenti riscontrati in tutti i Paesi europei, che però impattano in modo diverso a seconda dell'*energy mix.*

Rimane il punto per me fondamentale: non è accettabile questo incremento del prezzo del gas, che quindi è a monte di un'intera filiera che abbiamo poc'anzi discusso e che effettivamente si traduce solo nel risultato di una grande speculazione da parte di certi *hub* che non producono, ma fanno solo transazioni. Penso,

alle possibili misure per incrementare la sicurezza del sistema nel breve e medio termine, nel corso delle ultime settimane sono state attivate misure con impatto a breve e medio termine, anche con missioni nei Paesi produttori (Qatar, Algeria, Angola e Congo) - perché questa è la parte di diversificazione che si stima possano portare complessivamente a ridurre la dipendenza di circa 20 miliardi di metri cubi all'anno. Tra queste citiamo l'incremento delle importazioni di gas algerino. è ipotizzabile un incremento di 9 miliardi di metri cubi all'anno. Per questo è indispensabile un accordo con il Governo algerino, per ottenere forniture aggiuntive via gasdotto

l'incremento dell'*import* sull'infrastruttura Trans Adriatic pipeline (TAP): si può aumentare di 1,5 miliardi di metri cubi all'anno in tempi abbastanza rapidi, tramite interventi sulle centrali di spinta di Albania e Grecia, a patto di avere volumi aggiuntivi dall'Azerbaigian. punto è la massimizzazione di utilizzo dei terminali di gas naturale liquido. In particolare potremmo incrementare l'utilizzo dei terminali italiani anche nei periodi dell'anno in cui tipicamente non sono utilizzati, con un incremento possibile di circa 6 miliardi di metri cubi l'anno. Questo significa disponibilità di GNL aggiuntiva e un miglior utilizzo dei terminali, come per esempio recentemente discusso con il Qatar. C'è poi l'incentivazione dell'iniezione di gas in stoccaggio, per far sì che il ciclo di riempimento degli stoccaggi, che si sta avviando ora in previsione del prossimo periodo invernale, sia il più rapido ed efficace possibile, per garantire che le misure di risparmio di gas di cui sopra abbiano l'effetto di ottenere l'effettiva iniezione di gas in stoccaggio. Altrimenti, si ridurrebbero solo in un mero *import*. Sono tutti punti che vanno regolati con strumenti regolatori che sono in fase di valutazione.

abbiamo qualche mese di autonomia per produrre un po' più di elettricità. Ovviamente tutto quello che stiamo cercando di fare - e lo dico qui, che sia chiaro a tutti - a parità di gas, sperando non ci sia una

di misure in favore delle rinnovabili. In questi giorni state discutendo la conversione in legge del provvedimento che prevede la liberalizzazione sino a 200 chilowatt, che è tanto, delle rinnovabili come fossero manutenzioni. Abbiamo sbloccato mezzo gigawatt di impianti eolici pochi giorni fa. Stiamo cercando di accelerare, perché la via maestra rimane comunque sempre quella di ridurre i consumi, da un lato, e di accelerare le forme alternative che sono *greenhouse* *gas* *free*, dall'altro. Sempre pensando ai prossimi periodi invernali, oltre a quelle descritte, si potrebbe intervenire con misure di contingentamento della domanda e di accelerazione dell'efficientamento energetico, quindi misure di flessibilità sui consumi di gas (come l'interrompibilità del settore industriale, che però deve agire per brevi periodi settimanali, solo in caso di picchi della domanda), anche nel settore termoelettrico (dove pure esistono misure di riduzione del carico in modo controllato), e misure di contenimento dei consumi negli altri settori. c'è un piano di riserva di contenimento dei consumi a diversi livelli, a seconda del grado di emergenza. Sono cose pronte, lo Stato le ha e, se dovessero servire, verranno messe in atto. È chiaro che ci si prepara a tutti i possibili scenari, sperando che non si avverino quelli peggiori. Si può poi sempre pensare a un incremento di importazioni di energia elettrica dal Nord Europa per ridurre il consumo di gas nel parco termoelettrico italiano. Le possibili misure strutturali per eliminare invece la dipendenza totale di importazioni dalla Russia richiedono alcune riflessioni. Vi dico i punti fondamentali della strategia. È chiaro che qui è stata avviata una riflessione su misure strutturali che devono essere in linea con le proposte del pacchetto europeo che è in corso di finalizzazione, RePower EU: Joint european action for more affordable, secure and sustainable energy, che sta per uscire e prevede misure importanti. Stiamo valutando la nostra capacità di rigassificazione su unità galleggianti,

Per essere molto chiari, si tratta di navi che fanno rigassificazione vicino al punto di ingresso. Questa soluzione è rapida e flessibile rispetto a terminali *on-shore* fissi a terra ed è di minor costo, anche se - come potete capire - a livello europeo è partita la corsa alle navi di rigassificazione: non sono tante e costruirle richiede molto, quindi si devono prendere quelle che ci sono. Quanto ai costi di affitto elevati, per fortuna ci siamo mossi per primi, avendo l'idea della nostra dipendenza molto forte, e abbiamo ora due o tre opzioni che stiamo valutando. Nuova capacità di rigassificazione *on-shore*: in particolare, sono anche realizzabili progetti per terminali a terra, che potrebbero garantire circa 20 miliardi di metri cubi all'anno. di trentasei-quarantotto mesi, quindi sono infrastrutture un po' più grosse; intanto si può vedere l'evoluzione, avendo comunque quelli galleggianti che sono permanenti. permanenti. Le cose che vi ho detto però non sono cumulabili: l'idea non è di fare tutto, poiché sarebbe eccessivo e richiederebbe anche forniture di GNL molto forti, ma stiamo valutando in termini di tempi, di costi e di efficacia come arrivare ad avere

Tenete conto che questa seconda misura avrebbe bisogno anche di alcuni interventi in Albania e Grecia per le stazioni di pompaggio, quindi sarebbe un'operazione internazionale piuttosto complessa; però la stiamo analizzando.

ogni 8 gigawatt di potenza elettrica che installiamo ci fa risparmiare in media 3 miliardi di metri cubi di gas.

nel medio-lungo periodo non si vede il problema. Aggiungo che ci sono un incremento di produzione nazionale di 2,2 miliardi di metri cubi del nostro gas - questo l'abbiamo discusso di recente - dalle attuali stazioni di estrazione, che sarà

Ricordo inoltre l'annullamento transitorio degli oneri di sistema, il potenziamento del *bonus* sociale, la riduzione dell'IVA sul gas e l'introduzione di contributi straordinari sotto forma di credito d'imposta: sono le cose che avete visto nelle recenti misure. l'introduzione di interventi a favore del settore dell'autotrasporto, il sostegno alle esigenze di liquidità delle imprese e gli interventi sull'elettricità prodotta da impianti rinnovabili (che godevano di incentivo fisso pre-2010). È chiaro che, come vi dicevo poc'anzi, abbiamo avviato una fittissima discussione a livello europeo con la Commissione, proprio in vista del piano RePower EU. Tenete conto che la direttiva prevede misure per mitigare l'impatto sui prezzi residenziali e per piccole imprese, soprattutto a livello di *retail*; regole per aiuti di Stato che consentano di far fronte agli elevati costi energetici per le imprese; misure per la tassazione di extraprofitti per finanziare le misure di supporto. Questo lo prevede il piano RePower EU, quindi tutto quello che stiamo facendo adesso lo stiamo facendo con un occhio a RePower EU, che probabilmente uscirà

Il *price cap*, oltre a portare beneficio diretto ai consumatori di gas (perché si dice che l'Europa intera si dovrebbe presentare al mondo con un *price cap*),

Per venderne una quantità notevole come quella a cui stiamo pensando, bisognerebbe fare delle infrastrutture e occorre del tempo. In questo tempo noi ci attrezziamo con il nostro *energy mix* e con tutte le misure necessarie, per esempio le rinnovabili, il risparmio e i futuri *energy mix*, e avremo tempo di diventare più autonomi. La seconda misura che abbiamo proposto è il disaccoppiamento dei prezzi di vendita dell'energia prodotta dalle tecnologie rinnovabili rispetto alla produzione termoelettrica. Su questa cosa sono stato molto insistente;

adeguandomi al prezzo dell'energia termoelettrica prodotta con il gas? Questa misura è stata proposta tanti anni fa quando aveva senso perché la rinnovabile costava molto e il gas era molto economico e quindi serviva, grazie agli utili dello Stato, a incentivare l'uso della rinnovabile. Adesso, per una serie di motivi che abbiamo discusso anche con qualche perplessità, il gas costa troppo ed è doppiamente sbagliato agganciare le rinnovabili a quel valore di mercato. Quindi: *price cap* sul gas uguale per tutta l'Europa (sarebbe una grande notizia) e sganciamento del prezzo dell'elettricità dal prezzo del gas. Sembrano due cose ragionevoli, che ovviamente vanno a incidere enormemente su delle regole di mercato molto consolidate e complesse da cambiare. Concludo con l'andamento dei prezzi del carburante per autotrazione, che è l'ultimo nella catena: gas ed elettricità, parliamo di benzina e diesel. Per quanto riguarda il costo dei carburanti da trazione, dall'inizio dell'anno c'è stato un aumento dei costi del Brent che ha toccato punte di 130 dollari al barile, partendo da 78. Il valore del barile si attesta in questi giorni intorno a 100 dollari. Da questo conseguono in parte gli aumenti dei costi del carburante, che hanno suscitato anche apprensione da parte di numerose categorie produttive. Non dimenticate però quello che dicevamo prima: è proprio il costo dello stesso gas, della stessa energia, che serve nelle raffinerie a trasformare

cosa vado a memoria). Quindi, c'è un'oggettiva diminuzione della disponibilità di diesel. Sulla benzina il problema è meno rilevante dal punto di vista delle quantità. C'è un problema di mercato perché il costo del barile è aumentato e di costi della produzione di questi carburanti finiti che mettiamo nel serbatoio, che si lega a quanto vi ho detto in precedenza. Per mitigare l'incremento del Brent Stati Uniti e Unione europea hanno operato una *oil release*. Abbiamo aderito a questa proposta contribuendo con 2 milioni di barili nel periodo marzo-settembre,

Poiché c'è stato un maggior gettito IVA, dovuto al fatto che la base è aumentata, tale maggior gettito potrebbe essere utilizzato per ridurre l'accisa corrispondentemente e avere una diminuzione di prezzo alla pompa. Sappiamo benissimo che operare sui carburanti da trazione è molto complesso.

un po' di carenza di diesel e del costo in crescendo (veramente un po' esagerato, a questo punto) del gas e dell'energia che serve ai processi industriali. Mi fermo qua. Vi ringrazio per l'attenzione e spero che quanto vi ho detto sia chiaro.

ringraziamo lei, ringraziamo la Conferenza dei Presidenti di Gruppo e naturalmente ringraziamo il signor Ministro, perché pensiamo che su questo tema stiamo rischiando moltissimo. Nella vita quotidiana delle famiglie questa vicenda sta pesando come uno *tsunami*, sia per esigenze strettamente economiche che per una questione di fiducia. Dopo due anni di Covid, arriva una botta ulteriore; e sappiamo quanto sia importante la fiducia nell'economia. Dunque, abbiamo chiesto questo appuntamento e ci dichiariamo soddisfatti, signor Ministro, delle sue considerazioni. Aggiungiamo le nostre, molto brevemente; il tempo non permette altro che dei singoli *tweet*. Prima, però, premettiamo che stiamo parlando di una guerra e, quando si parla di una guerra, la prima immagine, il primo pensiero, il primo momento di riflessione vanno a quelle famiglie che stanno perdendo i propri cari, a quelle immagini delle donne incinte che perdono i bambini, a quelle immagini di famiglie che vengono costrette a lasciare l'Ucraina ribadendo che c'è un aggressore, la Russia di Putin, e c'è un aggredito, l'Ucraina. Su questo non ci possono essere dubbi. C'è un elemento in più, tuttavia; io penso che siamo in presenza di uno stravolgimento. Quelli che dicono che ciò che sta facendo Putin è umorale a mio giudizio sbagliano. Quello che sta facendo Putin è immorale, ma non è umorale; è figlio di una visione strategica che sta spostando a Est la mappa del mondo. Su questo ha ragione il signor Ministro a dire che ancora non ci sono i gasdotti; ma negli accordi del 2021 e del 2022 è evidente che c'è un patto Russia-Cina che si apre al Sud-Est e, più in generale,

quale missione strategica ha? Quella di combattere i terroristi islamici e i *cyber attack* o di essere un ricordo del passato? È un grande tema, di cui non possiamo discutere qui oggi. Quello che è certo è che il mondo si sta spostando a Est e che la Cina è sempre più centrale. Da questo dobbiamo partire. Per arrivare a dire cosa? Per arrivare a delle conseguenze nella nostra vita. Oggi, con quanto accaduto, grazie anche all'azione del Ministro, è evidente che è finito il tempo del no a prescindere sugli impianti. Per un quindicennio c'è stata una ubriacatura da no a prescindere. Io ho fatto il Presidente della Provincia e avevo i comitati del no ai termovalorizzatori. Ho fatto il sindaco e avevo il no per qualsiasi intervento sull'energia. Ho fatto il Presidente del Consiglio e avevo il no sul TAP. Ora non voglio stare a rivendicare quello che abbiamo fatto noi. Il punto fondamentale è che in questo pianeta o si pone il tema dell'energia come chiave, non soltanto per una questione economica, ma per una questione di giustizia, oppure ci portano tutti via e saremo sempre più insignificanti nello scacchiere internazionale che cercavo rapidamente di delineare. Per questo è assurdo che ci siano delle Regioni che hanno bloccato non solo le trivelle, ma le rinnovabili. E ciò è accaduto in questi mesi e bisogna avere il coraggio di dire che ha fatto male al nostro portafoglio e alla nostra credibilità. Dopodiché, signor Ministro, lei ha detto che porterà in Europa la proposta italiana perché ci sia un tetto ai costi ed è fondamentale, anche perché, se giustamente si dice che c'è una truffa - lei ha fatto bene a dirlo - è chiaro che i truffati sono i cittadini, ma bisogna anche dire con forza che i truffatori devono essere messi in condizione di non truffare più. Il punto fondamentale è che serve un tetto, perché la casa degli italiani ha bisogno di un tetto al costo della benzina e al costo delle bollette, che stanno facendo impazzire le nostre famiglie. Per concludere, saltando tutta una serie di considerazioni che avrei voluto farle, signor Ministro, va bene andare nella direzione di mettere un tetto finale alle spese degli italiani, però si abbia anche il coraggio di inserire questa dinamica in una cornice più ampia. Sta cambiando il mondo il mondo rende necessario un nuovo protagonismo dell'Italia. Non si può fare un ragionamento di lungo periodo senza pensare che nel frattempo le famiglie, le imprese, le RSA, il mondo delle scuole e della quotidianità stanno soffrendo una crisi che non era prevista e non ha paragoni immaginabili negli ultimi trent'anni. Buon lavoro, signor Ministro,

il Ministro per l'informativa che ci ha dato, anche perché vi sono

gas. Aggiungo che siamo di fronte ad una speculazione vera e propria. Lei, signor Ministro, ha affermato che c'è un aumento speculativo, ma quando ci sono gli aumenti speculativi

il costo di un barile Brent era di 147,50 dollari;

del gasolio ha superato quello delle benzine, arrivando a oltre 2,3 euro al litro, nel 2008

Per evitare la fiera dell'ipocrisia il Ministro ha affermato che bisogna fare le accise mobili. Io ho presentato decine di volte emendamenti al riguardo, abbiamo fatto conferenze stampa in sala Nassirya per le accise mobili e per fissare un tetto, ma purtroppo tutti quegli emendamenti sono stati bocciati, anche perché

«Le guerre - signor Presidente - sono fatte da persone che si uccidono senza conoscersi, per l'interesse di persone che si conoscono ma che non si uccidono», come scrisse il grande poeta cileno Pablo Neruda. Bisogna lavorare per soluzioni diplomatiche, non alimentando il conflitto con le armi. Signor Presidente, lavoriamo tutti per soluzioni diplomatiche e per la pace.

Questo Governo sarà ricordato nella storia italiana per l'assoluta incapacità di gestire e di risolvere i problemi. Avete cominciato con il *green pass*, strumento usato per costringere le persone a vaccinarsi, e lo tenete ancora in piedi, nonostante la pandemia sia finita in tutto il mondo. La crisi economica bussa alle porte delle nostre famiglie e delle nostre imprese e ancora vi ostinate a tenere i lavoratori senza *green pass* fuori dal lavoro, provocando un danno sia alle famiglie, sia all'economia. Veniamo al tema del caro energia e del caro bollette. Lei ha sostenuto che è in corso una truffa, ma i controllori dove sono? Il Governo dov'è? Dov'è super Mario Draghi, quello che ha messo insieme una maggioranza larghissima, tanto larga da non entrare neanche più in questo Parlamento e da buttare fuori il Parlamento stesso? L'uomo del *whatever it takes*, l'uomo che ha salvato l'euro, perché adesso non salva le famiglie? Forse perché per un banchiere centrale, che si è formato in Goldman Sachs, la finanza è più importante dell'economia reale, i mercati sono più importanti delle famiglie. La sua relazione non è stata per nulla convincente, Ministro. Alla fine, il messaggio che resiste, che resta appiccicato è quello per cui dobbiamo rassegnarci ad abbassare i termosifoni e a consumare meno energia. Le vostre scelte comporteranno sofferenza e chiusure. Avete scelto di partecipare a una guerra dando armi e strumenti militari ad una delle parti e ora vi stupite che il mercato reagisca, che il mercato sia posseduto dal demone del neoliberismo e quindi speculi. Specula più facilmente quando uno Stato non è sovrano. Oggi bloccate gli oneri di sistema, che è cosa diversa da un intervento strutturale di revisione sugli oneri di sistema. Nei mesi scorsi avevo più volte invitato il Parlamento e il Governo a riflettere sul fatto che si potesse premiare il consumatore che consuma energia rinnovabile, togliendo gli oneri sistema; con quegli oneri di sistema saremmo andati a incentivare le rinnovabili. Ma è rimasta lettera morta e, ancora oggi, quel principio è e rimane lettera morta. Non volete capire che bisogna intervenire in maniera strutturale. Le famiglie si accorgeranno di questo gioco di prestigio. Gli oneri di sistema aumenteranno nei prossimi trimestri, così come stanno tornando le cartelle esattoriali e tutte le scadenze che avevate sospeso e tenuto congelate, ma che ad un tratto si stanno scongelando.

Non c'è alcun intervento vero di investimento sulle rinnovabili e sulle politiche energetiche. Per smarcarci dalla Russia, voi andate in Qatar e in Azerbaijan, due noti campioni di democrazia:

ci ha riportato dati che in buona sostanza aveva già comunicato nei giorni passati nelle varie audizioni. Non solo la Russia è un problema per quanto riguarda l'approvvigionamento: ci sono

L'idea di avere un mercato separato per quanto riguarda le rinnovabili è un'idea che va implementata, soprattutto in questo momento, anche per ragioni di velocità, con contratti di lungo termine per le rinnovabili, in modo tale da avere dei prezzi garantiti

che sono stati bocciati e sono scomparsi dagli ultimi provvedimenti adottati, in particolare un fondo di garanzia per le imprese che vogliono autogenerare elettricità

stiamo girando l'Italia da due anni per informare sulle comunità energetiche, introdotte durante il Governo Conte e che sono ancora

Costruire impianti a fonti rinnovabili, in questo momento, è la soluzione più veloce e moltissimi italiani non si rendono conto che autoprodurre elettricità diventerà sempre di più un fattore distinguente, perché a parte

Il gas deve essere utilizzato per le industrie *hard to abate*, finché non avremo abbastanza idrogeno per cambiare anche quel settore, ma sulla mobilità e sulla logistica si deve spostare spostare una struttura intera, bisogna spingere moltissimo sul trasporto pubblico locale e sulla rotaia, che sono un sistema estremamente più efficiente e i risparmi che potremmo conseguire in tal senso

finestra") *(IV-PSI)*. Signor Ministro, onorevoli colleghi, oggi non parliamo soltanto, come ha fatto il ministro Cingolani, di misure strategiche per fronteggiare una straordinaria emergenza energetica. Discutiamo anche - questa è la richiesta avanzata dal Gruppo di cui faccio parte - di misure da assumere nell'immediato e di un nome e un cognome da dare alla colossale truffa alla quale l'Italia e in larga parte l'Europa hanno assistito. Tre anni fa, signor Ministro, presentai un'interrogazione che riguardava il costo dell'energia elettrica: nessuna risposta. Due anni fa ripresentai quell'interrogazione, sempre sullo stesso oggetto: nessuna risposta. Un mese fa - se ne convinca: non ho informazioni particolari che mi provengano da mondi, servizi segreti o altro o altro - ho depositato un'interrogazione dove già si parlava di extraprofitti nel mondo del gas; non era scoppiata alcuna guerra, Putin non aveva ancora invaso l'Ucraina, però la traccia era evidente. Ho apprezzato il suo coraggio quando ha parlato con la chiarezza che l'ha contraddistinta,

speculatori finanziari di questa natura, è cosa indicibile. Ora dobbiamo, però, avere il coraggio di fare un passo in più. Lei stamattina ha parlato giustamente di misure da assumere oggi e di una previsione strategica delle misure da assumere

tanto di nome, cognome e indirizzo - non vorrei insistere, ma hanno un nome, un cognome e un indirizzo anche i grandi speculatori finanziari. E poiché hanno un nome, un cognome e un indirizzo, quindi, una residenza, è possibile colpirli; è possibile colpire gli extraprofitti con normative comunitarie, naturalmente, soprattutto, ma è possibile e doveroso colpire anche gli extraprofittatori, che sono i pescecani di cui parlava Scalarini cent'anni fa. Vado al punto e concludo. Sappiamo benissimo, anche se la cosa è sconosciuta al 98 per cento degli italiani, i quali ritengono che l'aumento del prezzo del gas e dell'energia siano figli della guerra, solo in piccolissima parte è così; anzi, non è così. Non lo è. Il prezzo finale del gas - lo sappiamo - non dipende né dalla domanda né dall'offerta; l'aumento nasce perché sui contratti di acquisto e di vendita gravano scommesse fatte dagli operatori finanziari. Ci sono fondi - domando, anche italiani? ci sono banche - domando, anche italiane? - che scommettono sull'andamento di quel prezzo e, nella misura in cui scommettono che il prezzo risalga (causa anche conflitti geopolitici), il prezzo naturalmente risale, con diversi effetti. Ne ricordo due in aggiunta ai suoi. Il primo: siccome il prezzo di tutte le tipologie di energia è parametrato sul gas, come è noto, quando il prezzo del gas sale, cresce anche il prezzo delle rinnovabili e dell'energia. C'è dell'altro: cresce naturalmente il prezzo di altri prodotti. C'è dell'altro ancora: siccome l'inflazione per due terzi dipende dall'energia, tenendo sotto controllo il prezzo del gas, l'inflazione prevista oggi intorno al 5 per cento - dicono gli economisti - potrebbe calare attorno al 2. Non aggiungo altro. Non parlo delle misure; condivido le sue. Il senatore Renzi ha ricordato quali dovrebbero essere quelle a corredo di questa iniziativa, però - ho concluso, Presidente - non si fermi, Ministro; accerti perché a quelle interrogazioni i Governi precedenti a questo non hanno mai dato risposta. Capisco che si tocca un terreno molto scivoloso, forse anche con effetti nazionali, e non solo riferiti a *hub* planetari, marziani o addirittura di Plutone. No, io parlo di Italia. Quelle risposte le dobbiamo alle famiglie italiane e a chi si impegna nella crescita economica di questo straordinario Paese.

onorevole Ministro, ho ascoltato con attenzione ciò che lei è venuto a raccontarci in Aula e le dico che ho avuto l'impressione che la sua fosse una relazione, una lezione quasi da Università, spiegandoci i metri cubi, spiegandoci vari problemi, da dove importiamo il gas e altro. altro. Signor Ministro, credo invece che in quest'Aula, quella del Senato della Repubblica, lei oggi avrebbe dovuto portare delle soluzioni. Avrebbe dovuto far capire agli italiani cosa sarà della loro vita, delle loro imprese, delle loro famiglie nelle prossime settimane. Invece, di tutto questo non ha detto assolutamente niente. Secondo noi ci sono due elementi che sono fondamentali: la guerra che Putin ha scatenato all'Ucraina ha cambiato e sta cambiando il mondo.

Se non erro, circa il 40 per cento delle risorse sono sulla transizione ecologica. Lei pensa che in questo momento, dove stanno bombardando, dove stanno uccidendo, il tema sia la transizione ecologica o la sopravvivenza delle nostre industrie e delle nostre famiglie? Già quando è venuto in audizione in Commissione industria aveva giudicato la mia domanda provocatoria. Non è provocatoria, signor Ministro, ma semplicemente di buon senso. Nella vita, infatti, non tutto è un paracarro inamovibile. Se ci sono delle situazioni, che certamente nessuno di noi aveva messo in conto e che stiamo vivendo, le cose si cambiano. Siete il Governo dei migliori. C'è un Presidente del Consiglio sicuramente autorevole, che in Europa può esprimere, senza se e senza ma

reale. Tutto quello che è successo, infatti, ha sicuramente impattato moltissimo sulla nostra vita economica. Pertanto, è il momento di capire cosa bisogna fare.

per tranquillizzare tutti quei settori produttivi altamente energivori e forse farli lavorare più tranquillamente. Signor Ministro, allorquando voi immaginate, perché non abbiamo contezza di questo, di non intervenire sui prezzi o forse di intervenire tardi, buttando via il tempo, quel tempo che le imprese e le famiglie non hanno? Se voi non

licenzieranno ed il costo sugli ammortizzatori sociali sarà molto più alto rispetto all'intervento che oggi dovreste fare.

Ha visto cosa sta succedendo nel settore dei trasporti? Noi siamo uno dei Paesi con il più alto numero di camion per il trasporto su gomma e se si fermano loro, si fermerà tutto,

che l'energia è un bene primario. Fino ad ora, infatti, le ho parlato di aziende e di famiglie, ma potrei anche parlarle di tutte quelle persone disabili e fragili, che in questo momento sono attaccate a delle macchine per poter continuare a vivere.

speculatori, ci deve dire se sono delle persone fisiche, e in quel caso si deve dire nome e cognome, o se gli speculatori e i truffatori sono coloro che oggi determinano il prezzo,

lo afferma da molti giorni e ieri è stata anche presentata una mozione alla Camera. Le nostre proposte sono semplici ma efficaci e soprattutto impatterebbero domani sulla vita delle imprese e delle famiglie.

rilevava settimanalmente il prezzo medio dei carburanti e riportava un prezzo finito di 1,95 euro al litro per la benzina verde; come sappiamo, però, ha superato abbondantemente i 2,30 euro. Anche in

di angoscia e di imprese che rischiano di chiudere; anzi molte hanno già chiuso e altre stanno per chiudere a fronte dei rincari dell'energia.

La sicurezza energetica del nostro Paese, prezzi ed energia accessibili costituiscono questioni strategiche fondamentali per noi, per le imprese e le nostre famiglie.

vanno denunciati nomi e cognomi. Le magistrature hanno aperto dei filoni d'inchiesta, ma noi abbiamo la responsabilità politica, nel momento in cui denunciamo e facciamo bene a denunciare fatti del genere, di individuare i responsabili e, di conseguenza, di trovare i rimedi. Il Partito Democratico non è stato con le mani in mano e, proprio per affrontare gli insopportabili rincari delle bollette delle famiglie e delle imprese, ha proposto

alla riduzione delle accise, collegata alla sterilizzazione dell'IVA, al sostegno agli autotrasportatori, alle imprese energivore e gazivore cosiddette *hard to abate,* quelle cioè che consumano enormi quantità di energia per svolgere il proprio processo industriale

misure. Le nostre imprese vanno aiutate e salvaguardate perché escono dagli anni drammatici del Covid ed entrano in anni altrettanto drammatici a causa del costo dell'energia. Lo stesso impegno che il Governo ha messo nei due anni

una presentazione, anche molto analitica dal punto di vista quantitativo, che parla di milioni di famiglie che possono essere sostenute nel caro bollette nel corso delle prossime settimane e dei prossimi mesi. Come finanziare tutto ciò, Ministro? Certamente, nel momento in cui diciamo che ci sono degli extraprofitti, dobbiamo avere anche il coraggio di dire che tali profitti, che riguardano non la capacità manageriale delle imprese, imprese, ma condizioni esogene alle stesse, hanno comportato altri profitti o profitti utili per quelle imprese anche di miliardi di euro: a livello europeo 200 miliardi di euro nel 2021; a livello nazionale ci sono imprese che hanno avuto extraprofitti per centinaia di milioni di euro rispetto al 2019. Allora è giusto far sì che questa ricchezza, che non è dovuta a una capacità strategica manageriale, venga redistribuita a coloro che ne stanno pagando il prezzo, e quindi alle imprese e alle famiglie. *(Applausi)*. Il contributo di solidarietà per questi extraprofitti ci sembra, pertanto, un'operazione assolutamente da fare. Siamo molto felici - naturalmente non è merito nostro - di vedere che il nostro progetto, che aveva assunto addirittura la forma di un emendamento

È veramente strabiliante: siamo a 160 euro per megawattora; ma stiamo pensando di portarlo - nel progetto del presidente Draghi, se ho capito bene - a 100 euro il primo mese, per poi scendere a 90-80 euro.

perché i singoli Stati non sono in grado di gestire operazioni di questo tipo, per evidenti ragioni. Allo stesso modo, il disaccoppiamento dei prezzi di vendita tra energia rinnovabile e altre fonti deve essere certamente una grande azione del Governo nazionale, ma deve essere in collegamento con una grande azione a livello europeo. Signor Ministro, a tale riguardo appoggeremo pienamente il Governo perché sappiamo che questa è l'intenzione. Qui c'è il secondo passaggio e poi c'è il terzo: come riuscire a realizzare l'autonomia energetica nazionale e l'autonomia energetica dell'Unione europea? Il primo punto è eliminare o ridurre drasticamente la dipendenza dai gas e dal gas russo.

Siamo però contemporaneamente anche il secondo Paese in assoluto a livello europeo per il consumo dei gas nella produzione dell'energia totale, dopo l'Olanda.

anche perché, se spostiamo la nostra dipendenza energetica dall'instabilità russa all'instabilità algerina e congolese, è del tutto evidente che non è la risposta del futuro. Non so se mi spiego.

a meno che non vogliamo dipendere in futuro dai gas, ma sappiamo benissimo che le grandi riserve di gas a livello mondiale sono in Iran e in Russia, e con questo abbiamo già detto tutto. tutto. Vado al terzo passaggio, signor Ministro. L'autonomia energetica deve camminare su un binario più avanzato rispetto alla risposta immediata - quella del gas - che dobbiamo giustamente dare. Elettricità Futura, che rappresenta 500 aziende di Confindustria e il 70 per cento della produzione nazionale, ha presentato progetti per 60 gigawatt di energie rinnovabili da

80.000 posti di lavoro e l'equivalente energetico di un taglio di 15 miliardi di metri cubi di gas, e cioè più del 50 per cento dell'importazione nazionale dalla Russia. All'esito dell'ultima asta di Terna nel mercato delle capacità, Enel ha deciso di non convertire nemmeno a gas le centrali di La Spezia, Civitavecchia e Brindisi.

Nel lungo periodo è di ogni evidenza che è conveniente economicamente, socialmente e politicamente per il nostro Paese continuare con grande determinazione lungo tale strada. Su questo il Governo avrà il nostro appoggio. *(Applausi)*.

e lo invito subito, in premessa, a non lasciarsi intimorire dalle polemiche che ci sono state quando ha giustamente parlato di speculazione.

termine. Cosa è accaduto? Qualcuno qui, all'inizio di questa discussione, parlava del fatto che i soliti bloccavano le rinnovabili. Ma i dati sono chiari: dal 2014 purtroppo nel nostro Paese

della mobilità, per esempio. Noi siamo il Paese che credo abbia il *record* di trasporto delle merci su gomma. Faccio questo esempio per dire che, evidentemente, dobbiamo colmare oggi

È assolutamente importante quello che lei ha detto a proposito del tetto, del *price cap* a livello europeo. Ed è altrettanto, se non ancora più importante, il disaccoppiamento: noi siamo assolutamente d'accordo per quanto riguarda il disaccoppiamento delle rinnovabili rispetto

lo hanno già detto in tanti ed è sotto gli occhi di tutti: il mondo sta cambiando. È normale che il mondo cambi, ma lo sta facendo a una velocità incontrollabile e c'è bisogno di misure straordinarie, di una rivoluzione virtuosa come solo una grande crisi di sistema può produrre. La prima rivoluzione sarebbe riuscire a fermare la guerra. Stiamo Stiamo affrontando una pandemia globale, stiamo entrando in un'economia di guerra, anche senza carri armati sui territori, e ora c'è bisogno di grandi e veloci contromisure per non essere travolti. C'è bisogno di visione e di strategia, oltre che di tattica sull'emergenza. C'è bisogno di un'immediata, decisa e profonda azione di revisione dei sistemi in campo economico, finanziario, energetico e di conseguenza sociale. Via steccati e via muri ideologici che frenano le iniziative, nella consapevolezza che non abbiamo più tempo per sbagliare. *(Applausi)*. Il Paese va ascoltato seriamente per fargli ritrovare quella fiducia nelle istituzioni e nella rappresentanza democratica, della cui realizzazione siamo responsabili. Le famiglie e le imprese sono ormai - verrebbe da dire - alla canna del gas, ma non c'è né di gas,

lo può governare, grazie alla materia prima più preziosa e abbondante che questo Paese possiede, che è l'ingegno. *(Applausi)*. All'ingegno si aggiunge la grande capacità di intrapresa a ogni livello: dalla più piccola impresa artigiana alla più grande industria, questo Paese è in grado di compiere miracoli, se vengono però create le giuste condizioni. le giuste condizioni. L'Italia è un Paese che lavora e ha messo il lavoro tra i suoi valori fondativi, ma dobbiamo consentirgli di potersi muovere. Approfitto dell'occasione per ricordare Marco Biagi nella settimana dell'anniversario della sua morte. Ministro Cingolani, oggi con volontà propositiva Forza Italia, forza di maggioranza che sostiene il Governo, si rivolge a lei che può determinare le scelte sui temi più importanti in questo momento: energia, innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale, economica e sociale, concessioni, autorizzazioni, verifiche, controlli e sistemi di protezione. Oggi siamo al suo fianco per aiutarla a realizzare la trasformazione che il Paese si aspetta e che ha bisogno di tanto coraggio. Penso che a lei il coraggio non manchi, come non manca a noi che siamo qua oggi con lei, mettendo a terra una politica energetica che per trent'anni non è stata realizzata. Penso al PNIEC, al Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, già obsoleto e non ancora aggiornato. Semplifichiamo subito procedure, *iter* autorizzativi; incoraggiamo investimenti; premiamo e agevoliamo riconversioni riconversioni e innovazione delle imprese; rendiamo flessibile il lavoro puntiamo sulle comunità energetiche e sull'autoconsumo; rimettiamo in funzione le trivelle inutilizzate e usiamo il nostro gas subito. Diamo certezze a chi produce e crea lavoro con provvedimenti e incentivi strutturali, perché le aziende hanno bisogno di strutturalità, rendendo strutturale *in primis* il *golden power* almeno sul piano energetico; mettendo in sicurezza la salvaguardia dei nostri *asset* strategici come l'idroelettrico e le rinnovabili; prorogando le concessioni ai nostri operatori italiani per consentire loro nuovi investimenti e *revamping*; attuando il sacrosanto principio di reciprocità sia all'interno della Comunità europea, sia a chi viene da fuori, con lo Stato alleato delle Regioni che regolamentano. Poi, l'azione più importante: realizzare impianti in ogni punto d'Italia per potenziare la raccolta, lo smaltimento e il riciclo dei rifiuti. *(Applausi)*. I rifiuti sono un patrimonio. potenziare oltre misura l'economia circolare per poter produrre e utilizzare quelle materie prime seconde che possono sopperire la mancanza di materie prime. Ripeto: abbattiamo i muri ideologici. Basta con i comitati del «no», che dicono «no» persino alla realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile, pena una dipendenza che sta finanziando la guerra. *(Applausi)*. Questa dipendenza sta finanziando la guerra. Bisogna invece potenziare la formazione e le competenze per governare l'innovazione e informare correttamente i cittadini per superare quella sindrome di NIMBY che crea lo stimolo a volere fortemente la sostenibilità, ma sempre lontano dalla propria visuale, perché questa si chiama ipocrisia. Bisogna correre con i decreti *end of waste*; agevoliamo, velocizziamo, semplifichiamo le pratiche per il riciclo. Pensiamo alla produzione di residui; interveniamo sui consorzi, affinché agevolino. Non mandiamo più all'estero i rifiuti. Non paghiamo più per esportare valore

succedono queste cose. Facciamo correre la ricerca sul nucleare pulito. Facciamola correre, insegnando la differenza tra fissione e fusione; ricordando che non abbassiamo le tasse anche perché siamo già in infrazione per il deposito unico nucleare e perché paghiamo a caro prezzo l'esportazione dei nostri dei nostri rifiuti radioattivi. *(Applausi)*. Ministro Cingolani, lei è una persona preparata, schietta, diretta, che ha il coraggio di denunciare i problemi, che però bisogna risolvere. Noi oggi vogliamo suggerirle una rosa di soluzioni, che andrebbero attuate tutte insieme, subito. Lei che guida un Ministero assolutamente centrale nelle scelte ha una grande responsabilità e non abbia timore di condividerla con il Parlamento, voce del Paese, Paese, con le scelte e con la responsabilità. Siamo consapevoli che ci sarà da lavorare sodo subito, da lavorare duro non solo per tenere l'Italia a galla, ma anche per farla navigare e renderla finalmente libera e indipendente. Per questo bisogna innanzitutto dare risposte alle famiglie e alle imprese, preoccuparsi di farle sopravvivere oggi, per poterle poi portare a regime. Non bisogna aver paura. Bisogna stringere alleanze con chi produce e crea lavoro, con chi ha dimostrato di saperci fare, e lasciarlo fare, mettendosi al fianco fianco come facilitatori, stabilendo regole certe e sanzioni pesantissime per chi non le rispetta. Ci sono emergenze oggi e bisogna risolverle subito, a partire dal caro bollette e dal costo dei carburanti, la cui metà del prezzo è prelievo fiscale, che sta mettendo in ginocchio l'autotrasporto e a rischio gli approvvigionamenti. Se si ferma l'autotrasporto, si ferma il Paese, si ferma il commercio, si fermano gli ospedali, si fermano le scuole:

Togliere le accise è un investimento, non una mancata entrata. *(Applausi)*. Lo chiediamo con forza, lo stiamo chiedendo: costerebbe di più l'inerzia. Se si ferma l'autotrasporto, si ferma il Paese. Costano di più i 4 miliardi di truffe sugli eco *bonus* che non fermare gli speculatori, imponendo un tetto sui prezzi. Sono 200.000 le imprese in difficoltà; un milione i posti di lavoro a rischio, fornitori che non consegnano: non è uno scherzo. Rivediamo tutto ciò che ha dimostrato di non funzionare, rivedendo anche - e concludo - l'utilizzo del PNRR, aggiornando i progetti al periodo che stiamo vivendo. Non siamo nel 2019, non siamo nel 2020, non siamo nel 2021: siamo nel 2022 ed è successo

Nel 2001 l'Italia estraeva dai giacimenti nazionali 15 miliardi di metri cubi di gas, che rappresentavano il 15 per cento dei consumi totali, che allora erano 71 miliardi. Importavamo dalla Russia 20 miliardi di metri cubi, pari al 28 per cento del totale. Vent'anni dopo, nel 2021, lo scorso anno, il gas a chilometro zero estratto si è ridotto a 3,3 miliardi, il 4 per cento dei consumi totali, che nel frattempo sono saliti a 76 miliardi, e lo scorso anno abbiamo importato dalla Russia 29 miliardi di metri cubi, pari al 38 per cento In questi dati si riassume il fallimento di anni della politica italiana ed europea in materia energetica, impostata sul no a tutto. Non bastava il no al nucleare: si è aggiunto il no subito al carbone, il no alle trivelle, il no al TAP, il no ai rigassificatori, il no persino alle biomasse e alla geotermia. La politica nel nostro Paese, intrisa di ideologismo ambientalista, ha ignorato i fondamentali. Irresponsabilmente, in vent'anni si è alzata la dipendenza energetica estera del gas, passando dall'85 per Invece di diversificare gli approvvigionamenti, abbiamo fatto il contrario, incrementando le importazioni di gas russo. Inoltre, hanno prevalso in Italia, come in Europa, i fautori del *green deal*,

I fautori della transizione ecologica senza i fossili non fanno però alcuna distinzione tra olio combustibile, carbone e gas, che invece tra i fossili è quello meno inquinante. E così per le infrastrutture del gas da diversi anni si sono bloccati gli investimenti, estrazioni e rigassificatori. Fino a pochi mesi fa anche in Senato, da diverse forze politiche, il gas veniva considerato il male assoluto, mentre sta esercitando il suo ruolo strategico di accompagnamento alla transizione ecologica. Eppure, che si sarebbe andati a sbattere contro il caro bollette qualcuno l'aveva paventato a tempo debito: la Lega, al Copasir, già nel settembre 2020, chiedendo e ottenendo un'indagine conoscitiva sul sistema energetico; sempre la Lega, durante la predisposizione delle linee generali del PNRR. Cito le nostre osservazioni confluite nella relazione finale sulla proposta del PNRR approvata qui in Senato nel marzo 2021. marzo 2021. In un passaggio, in ordine allo sviluppo delle rinnovabili, si invitava il Governo a tenere conto dei seguenti obiettivi: «ridurre la dipendenza del Paese in termini sia di energia, sia di materie prime e diversificare le fonti di approvvigionamento; ridurre il costo delle bollette di energia elettrica e gas; rafforzare la sicurezza e la resilienza del sistema energetico del Paese con riferimento agli impianti, alle reti e alle riserve strategiche». Appelli evidentemente caduti nel vuoto. Ora, invece, parlano tutti di autonomia energetica, di diversificazione degli approvvigionamenti, dopo che il caro energia si è abbattuto come uno *tsunami* che sta travolgendo tutti e che rischia di vanificare la ripresa economica. Rispetto allo scorso anno, siamo a prezzi folli di elettricità e gas, che sono aumentati di sei volte. Il caro energia, che sempre più ha caratteristiche strutturali, è un fenomeno soprattutto europeo, ma l'Italia soffre molto di più perché paga le scelte discutibili di cui ho detto e per un *mix* energetico troppo ridotto. Ricordo come solo lo scorso anno il prezzo medio dell'energia elettrica in Italia è stato superiore del 30 per cento rispetto alla Germania e del 15 per cento rispetto alla Francia. Diamo atto al Governo di essere intervenuto negli ultimi mesi con cinque provvedimenti, stanziando oltre 17 miliardi per contenere le bollette di luce e gas fino al secondo trimestre di quest'anno. Ma le misure non sono sufficienti; la situazione è insostenibile per molte imprese. Occorre fare molto di più: uno scostamento di bilancio è ormai indifferibile. Intanto, l'Europa, dopo la guerra russo-ucraina, per fronteggiare il caro energia ha aggiornato la cassetta degli attrezzi dopo quella mezza vuota di ottobre. La Commissione ha presentato il RePower EU. sono apprezzabili, altre non ci convincono, ma meglio tardi che mai. Va bene l'inserimento di gas e nucleare nella tassonomia. va bene il riconoscimento del ruolo del gas nella transizione. Ora si parla non più di affrancamento dell'Europa dal gas, ma di affrancamento dal gas russo. Sono i progressi del pragmatismo. *(Applausi)*. Occorre stare attenti ad accelerare troppo la transizione all'energia pulita con prevalenza di rinnovabili; fotovoltaico ed eolico non sono programmabili, perché producono solo quando ci sono sole e vento, e rappresentano un forte limite alla sicurezza del sistema energetico, e i sistemi di accumulo sono lungi dall'essere tecnologicamente pronti, sviluppati e distribuiti sul territorio. Sono preoccupato per la stabilità del sistema energetico in Sardegna, dove l'asta del Capacity market è stata assegnata a un accumulatore di 500 Le ricette del Governo per l'emergenza gas sono positive: sia le misure per incrementare la sicurezza a breve termine sia quelle per ridurre ed eliminare la dipendenza di importazioni dalla Russia, come quelle che lei ha indicato prima. Ministro, contrasti la speculazione e persegua il prelievo se ci sono extraprofitti del gas, come già fatto per gli impianti a fonti rinnovabili. rinnovabili. Come Lega - sempre attenta ai temi del caro energia o della sicurezza del sistema energetico - chiediamo a lei e al Governo di fare di più: ribadisco la necessità di un significativo scostamento di bilancio per contenere il caro bollette. Non basta Non basta estrarre più gas dai soli giacimenti autorizzati. Sappiamo che c'è il Pitesai con troppi vincoli, ma non possiamo continuare a regalare il nostro gas alla Croazia o alla Grecia. Dobbiamo ricercare nuovi giacimenti di gas a chilometro zero per aumentare la nostra autonomia energetica, anche per tutelare l'ambiente *(Applausi)*, visto che con quello di importazione che con quello di importazione emettiamo molte più sostanze climalteranti. Per la diversificazione degli approvvigionamenti riprendiamo il progetto del gasdotto EastMed, in grado di portare in Italia gas naturale da Israele. Allarghiamo il *mix* energetico a tutte le rinnovabili. Occorre sviluppare non solo fotovoltaico ed eolico - hanno forti limiti di programmabilità - ma anche il geotermico, le biomasse e soprattutto l'idroelettrico l'idroelettrico *(Applausi)*, che ha bisogno di investimenti attraverso manifestazioni di interesse pubblico, e non di semplici proroghe che verrebbero per la terza volta impallinate dalla Corte costituzionale. Occorre più autonomia tecnologica: non chiudiamoci allo sviluppo del nucleare di ultima generazione pulito e sicuro. Occorre aprire un dibattito serio, scientifico e senza pregiudizi sull'energia dell'atomo e riaprire la ricerca sulla fissione. Se al 2050 vogliamo contrastare seriamente i cambiamenti climatici e ridurre a zero le emissioni di CO2; se vogliamo rispondere alla domanda crescente di elettrificazione; se dovremo erogare energia in modo stabile e continuativo e se vorremo produrre idrogeno a bassissime emissioni per superare il gas, sappiate - cari colleghi - che la tecnologia nucleare è l'unica che potrà consentirlo. Ora occorre anche fronteggiare il caro carburanti, caro Ministro. Come se non bastasse il caro energia, la crisi in Ucraina sta aggravando il caro carburanti che rappresenta un ulteriore *shock* energetico. La situazione critica sui mercati internazionali delle materie prime ha spinto al rialzo i prezzi della benzina e del gasolio che, da diversi giorni, hanno superato i 2,3 euro al litro. Con questi prezzi insostenibili si mette in crisi il settore dell'autotrasporto; si determina il blocco di numerose attività produttive; si determinerà un'ulteriore impennata dei prezzi di dettaglio per molti prodotti di largo consumo, creando un pesantissimo danno all'economia del nostro Paese. È indubbio che questi prezzi stanno determinando un significativo extragettito per le casse dello Stato, stimato quest'anno in oltre 2 miliardi di euro. A questo punto diventa necessario - e la Lega ha depositato una mozione che il Governo agisca come fatto da altri Paesi europei, quali la Francia, l'Irlanda, il Belgio e la Polonia, che hanno deliberato misure di restituzione degli extraintroiti fiscali portando immediati benefici alla cittadinanza. Chiediamo con forza, qui in Parlamento e in centinaia di Consigli comunali, di intervenire con una misura di urgenza, temporanea, per la non applicazione dell'accisa, magari secondo il criterio della cosiddetta accisa mobile, oppure introducendo un'aliquota di IVA ridotta sul carburante. Cingolani, quest'azione, che non necessita di coperture economiche, è necessaria per la tenuta del sistema economico dell'intero Paese: attuatela! Ministro, accolga queste proposte e la piena disponibilità della Lega alla collaborazione. Buon lavoro!

ma speravo che ponesse di più l'accento sulle speculazioni. Invece, in realtà vi ha fatto solo un accenno. Va bene lo stesso. A noi va bene, ma dobbiamo veramente accendere un faro su ciò che sta succedendo oggi. Colleghi, ammetto che, pur avendo delle nozioni tecniche, ieri sera brancolavo un po' nel buio nel parlare di tariffe dell'energia.

nelle bollette elettriche, per quanto riguarda il mercato tutelato, che rappresenta la maggior parte delle utenze in Italia, il prezzo è fatto grazie a delle regole, stabilite dalla legge e applicate da ARERA;

Finita la pandemia, tutti hanno iniziato a produrre, tutti hanno avuto bisogno di energia e la quotazione è schizzata in alto. Quindi, il valore è molto alto, tanto che è decuplicato il valore della quotazione internazionale,

l'Istat, che, grazie alla banca dati Coeweb, ci illustra il fatto che il prezzo dell'importazione del gas è nettamente inferiore rispetto alla quotazione TTF.

Quindi, bisogna prendere delle misure, ma bisogna intervenire adesso. Perché adesso? Perché l'ultima delibera dell'ARERA è del 30 dicembre 2021. La prossima arriverà il 30 marzo e, se non interveniamo entro quella data, le bollette dei prossimi mesi saranno

gas. In più produce anche il gas. Lei stesso, signor Ministro, ha detto che il costo di produzione del gas è molto basso. Quindi, qualche sospetto mi viene, ma sto parlando di sospetti. Se poi guardo gli utili di ENI, trovo che nel 2020 ha realizzato 1,9 miliardi di utili e nel 2021 9,67 miliardi di utili. qualche sospetto ce l'ho. Magari anche noi, come Stato, potremmo fare qualcosa, visto che l'ENI è una partecipata pubblica. Davvero, però, facciamo il possibile per intervenire sulle regole che stabiliscono il prezzo della bolletta. Se ha senso intervenire per riparare i danni

facciamo in modo che questo non avvenga. Facciamo in modo che la transizione ecologica continui. Continuiamo quindi a investire sulle rinnovabili, come lei sta facendo - apprezziamo il suo lavoro sul PNRR - ma cerchiamo di fare veramente il possibile affinché vengano tutelate anche le comunità energetiche, su cui noi del MoVimento 5 Stelle Bisogna fare il possibile per raggiungere la transizione ecologica apportando meno danni possibile. Pertanto, se il carbone è necessario adesso perché ora abbiamo bisogno di energia, è possibile intervenire, ma deve essere un'azione molto limitata nel tempo. Proteggiamo le rinnovabili. Proteggiamo il nostro Paese.

in sede referente ed approvato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022 n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, di salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19,

Presidente, suddivideremo l'intervento con i relatori Misiani e Damiani e con il relatore di minoranza Calandrini.

dell'emendamento del Governo riferito al decreto-legge n. 13 del 2022, e poi di tutta la parte emendativa in Commissione. È stato un lavoro importante dal punto di vista del merito e degli interventi posti in essere, quindi vale la pena

desidera trasmettere l'idea di un Parlamento non al passo con i tempi, i drammatici eventi bellici e il preoccupante scenario economico da affrontare. Per via di queste considerazioni, va

è una prima parte di un trittico di interventi che il Governo e il Parlamento stanno ponendo in essere insieme per riposizionare Italia nel nuovo contesto geopolitico e sostenere famiglie, imprese ed enti territoriali in questa transizione non solo energetica, che è forse la più difficile e dolorosa dalla Seconda guerra mondiale a oggi.

norme importanti per fronteggiare la prima fase della crisi energetica. Ci sono norme importanti per il primo trimestre del 2022

come le questioni del caro energia e caro carburante. Sono previsti interventi per oltre 80 miliardi di euro, che abbiamo chiesto in Senato e che il Governo ha recepito nel cosiddetto decreto energia, per far fronte e dare una prima risposta alla crisi del settore degli autotrasporti e della distribuzione.

Tuttavia, è assai chiaro a tutti noi sin da oggi che sia il decreto sostegno-*ter*, che quello energia, per quanto importanti, non saranno sufficienti per far fronte alla grave crisi energetica alla grave crisi energetica ed economica connessa anche alla difficoltà di approvvigionamento, al caro prezzi e alla conseguente dinamica inflattiva, creando un deciso problema di scenario

un terzo decreto che sarà davvero importante e di cui abbiamo parlato questa mattina anche con il ministro Cingolani, che prende le mosse dal *summit* di Versailles e verrà pensato nel Consiglio europeo dei prossimi allo studio misure come il tetto sul caro energia, il sostegno alle famiglie e alle grandi imprese energivore, ma anche a tutte le imprese fortemente esposte in termini di liquidità. È allo studio ed è fortemente spinta dal punto di vista politico dal Senato e dall'ordine del giorno di maggioranza una riscrittura del Temporary framework.

La maggioranza ha sigillato queste importanti norme e questa importante evoluzione di scenario e di risposta allo scenario in un ordine del giorno, che è nato grazie

Ringrazio anche il MEF, rappresentato della sottosegretaria Guerra, e ringrazio la sottosegretaria Sartore; hanno sempre dimostrato grande competenza, ma in questa in questa fase di conversione

particolarmente importante. Il lavoro di tutte le forze di maggioranza e anche delle forze di opposizione è stato costruttivo, serio, di qualità. I senatori hanno arricchito di grande consapevolezza la conversione di questo decreto-legge, cercando sempre la mediazione. la mediazione. Non era scontato, nemmeno in un momento così grave; però l'obiettivo di non disunire la maggioranza ha prevalso su ogni altro tipo di considerazione. Oltre ai contenuti, che sono stati di qualità, questo scrive un nuovo metodo il quale si possono abitare le istituzioni, specialmente in un grave momento di crisi come quello attuale. Signor Presidente, anche io mi soffermerò molto velocemente sul provvedimento e cercherò anche io di fare qualche passaggio politico, perché ritengo che - come appena detto la correlatrice Donatella Conzatti - stiamo approvando un provvedimento che sconta - ahimè un passaggio un po' diverso rispetto a un mese e mezzo fa. Abbiamo uno scenario politico ed economico completamente differente. Questo provvedimento era stato pensato politicamente da questa maggioranza e dal nostro Governo per uscire

esplicare le nostre proposte; invece non ci sono state o sono state poche e pertanto abbiamo dovuto cambiare impostazione. Tant'è che poi sono arrivati altri

Siamo stati sostenitori anche noi, nella manovra finanziaria, di un aiuto concreto ai commercianti e ai ristoratori per il sostegno all'occupazione del suolo pubblico, la TOSAP; a questo abbiamo trovato risposte perché anche nel milleproroghe c'è stata, senza oneri, la proroga delle autorizzazioni. Ci sono state queste risposte. Abbiamo insistito tanto, tutti insieme, e abbiamo condiviso con le opposizioni la possibilità in un momento del genere di dare sostegno e respiro alle famiglie e alle imprese con la riapertura dei termini della rottamazione-*ter* e ci siamo riusciti, perché la volontà politica di tutti noi è stata proprio di andare in questa direzione: il merito va a tutta la maggioranza e all'opposizione che ha sostenuto e ha voluto dal Governo

sui mutui. Questo è un altro problema che sta tenendo banco, soprattutto per le imprese, in un momento di difficoltà dovuto ai costi dell'energia, in cui un'impresa deve decidere, nel momento in cui si ritrova con delle bollette da pagare, se non accendere più la luce, non accendere più i forni (essendo quindi costretta a chiudere), oppure se pagare le rate dei mutui; o l'una o l'altra cosa, non si può fare diversamente. Allora

perché oggi è importante dare maggiore respiro e concedere un'ulteriore proroga. Il rafforzamento patrimoniale delle imprese è un'altra questione importante. Questi sono tutti temi, come dicevamo, politici, che siamo riusciti a mettere insieme per dare respiro a questo provvedimento e dare anche un senso politico e un indirizzo, che poi concretizziamo anche con l'ordine del giorno vincolante per il Governo, che mi auguro

delle nostre attività economiche si sono fermati; valutiamo adesso, nel momento in cui abbiamo risbloccato la cessione dei crediti, se vi è la possibilità

Signor Presidente, mi associo al ringraziamento che i miei colleghi relatori hanno espresso nei confronti dei Gruppi parlamentari di maggioranza e di opposizione e dei rappresentanti del Governo (saluto anch'io la sottosegretaria Guerra) per la qualità del dibattito e per lo spirito costruttivo con cui sono state condotte una discussione e una votazione degli emendamenti non semplici, perché le condizioni di partenza, come hanno ricordato i miei colleghi, erano molto complicate: una dotazione pressoché simbolica di risorse e tempi, nella fase finale, oggettivamente stretti. Nonostante queste difficili condizioni di partenza, credo che il Senato abbia fatto la sua parte fino in fondo nel lavoro di miglioramento del testo iniziale, con l'approvazione di circa 90 emendamenti, quasi tutti ordinamentali, ma in non pochi casi significativi e concretamente utili ai cittadini. Penso all'estensione dei codici Ateco interessati dall'articolo 7, all'esenzione dal pagamento dell'IMU per gli immobili inagibili nelle zone terremotate, alla rimessione in termini, alla rottamazione, al saldo e stralcio e a tanti altri emendamenti molto specifici, ma molto attesi da tante categorie di cittadini e di imprese. Noi avremmo voluto, signor Presidente, modificare molto di più, anche gli articoli 16 e 28, che peraltro sono stati riscritti dal Governo con un decreto-legge intervenuto successivamente al sostegni-*ter*;

Il tema a fine gennaio era sostenere le attività economiche penalizzate dalle restrizioni anti-Covid e affrontare i primi aumenti dei prezzi dell'energia; la guerra ha cambiato tutto e l'accelerazione indotta da eventi di portata storica che hanno sconvolto l'Europa e il mondo apre una fase drammaticamente nuova e deve portarci a ripensare tante nostre strategie, tante nostre scelte. In questi mesi il Governo ha messo in campo interventi importanti e molte risorse per fronteggiare l'aumento dei prezzi energetici, come ha ricordato anche oggi il ministro Cingolani: 16 miliardi di euro per finanziare tanti interventi, molti dei quali contenuti nel decreto-legge sostegni-*ter*, dall'annullamento degli oneri di sistema, al potenziamento dei *bonus* sociali, elettrico e gas, al credito d'imposta per gli energivori, al meccanismo di compensazione a due vie per i produttori di energie dal 24 febbraio l'invasione russa dell'Ucraina ha segnato una nettissima discontinuità e la crisi energetica, che già prima dovevamo fronteggiare, oggi ha assunto una valenza di sicurezza nazionale. L'obiettivo di sostenere le famiglie e le imprese - che rimane e, anzi, si intensifica - deve andare di pari passo con gli obiettivi dell'indipendenza energetica dell'Italia e dell'Europa, del nostro affrancamento dalle forniture di gas naturale, dell'accelerazione del processo di decarbonizzazione e di sviluppo delle fonti rinnovabili. La decarbonizzazione, che è fondamentale per contrastare il cambiamento climatico, si deve intrecciare con le misure da mettere in campo per fronteggiare l'emergenza. Tutto questo richiede un salto di scala nelle politiche del Governo. Ne abbiamo parlato giusto questa mattina, nel dibattito sulle comunicazioni del ministro Cingolani, e ne abbiamo parlato nel corso della discussione parlamentare sul decreto-legge sostegni-*ter*. Noi ci auguriamo che le proposte di cui si è discusso in Commissione bilancio e, da ultimo, questa mattina in Assemblea, vengano raccolte dal Governo e tradotte in tempi brevi, anzi brevissimi, perché la sofferenza delle famiglie e delle imprese è reale, molto severa e merita risposte in provvedimenti concreti, che siano all'altezza dell'emergenza senza precedenti che l'Europa e l'Italia sono chiamate a fronteggiare.

Signor Presidente, mi unisco ai ringraziamenti dei relatori di maggioranza al presidente Pesco, che devo dire ha sempre usato molta attenzione, nel lavoro della

Hanno ragione i relatori quando dicono che questo decreto di fatto è superato dagli eventi, ma voglio ricordare che il provvedimento era già insufficiente

spiccioli se consideriamo che questo comparto ha cessato la propria attività praticamente da quasi due anni, riaprendo con limitazioni solo nei mesi estivi e brevemente prima dell'ultima ondata di pandemia, che le ha viste restare chiuse fino ad un mese fa. Il settore calcola perdite pari a 1,2 miliardi di euro e ha visto decine e centinaia di imprese arrendersi, chiudendo le proprie attività. Bastano questi numeri a comprendere perché le risorse siano completamente insufficienti. altro settore in ginocchio è il turismo, a cui l'articolo 4 destina un incremento di 100 milioni di euro nel Fondo nazionale del turismo, che è stato istituito con l'ultima legge di bilancio. Tale fondo era dotato di 280 milioni di euro,

stesso discorso vale per il fondo da 200 milioni per il rilancio delle attività economiche e di commercio al dettaglio, anche questa una cifra largamente insufficiente per aiutare un settore che registra ancora un ammanco di 1,7 miliardi di euro per tornare ai livelli pre-pandemia.

Le statistiche ci dicono oggi che il prezzo del gas è aumentato di oltre il 600 per cento rispetto al 2020, similmente ha fatto il prezzo dell'energia elettrica al netto di questo il provvedimento che esaminiamo si limita a concedere agevolazioni alle imprese energivore, anche queste insufficienti, dando invece benefici limitati a tante piccole e medie imprese che pure risentiranno del caro energia. Manca, a nostro parere, in questo decreto, una visione strutturale per risolvere il problema, perché serve un intervento imponente da parte dell'Europa; dobbiamo ragionare in termini di scostamenti e questo Governo ancora non è convinto, non ne parla e il presidente Draghi continua a nicchiare su questo aspetto. Serve un nuovo *recovery fund*, perché se non si va in questa direzione, noi da soli non riusciremo a dare soluzione a questi problemi, quanto manca la coscienza di aver posto in essere politiche energetiche fallimentari, che sono state fatte in nome di un ambientalismo estremo e di un no a prescindere a qualsiasi impianto. Abbiamo portato l'Italia a dipendere totalmente dall'estero per i suoi approvvigionamenti. L'approccio contenuto in questo decreto-legge è del tutto temporaneo e volto a tamponare solo parzialmente un'emergenza che, come dicevo prima, è esplosa prima delle tensioni tra Russia e Ucraina ed è chiaramente destinata ad aggravarsi con il conflitto in corso. Confindustria stima che dal 2019 al 2021 il costo dell'energia per la manifattura sia passato da 8 miliardi nel 2019 a 21 nel 2021, fino a 37 miliardi nel 2022. Di fronte a questi numeri, analisi della CGIA di Mestre rilevano che gli interventi di questo decreto-legge coprono solo il 6 per cento di tutti gli aumenti che si sono verificati, che nel frattempo mettono a rischio 500.000 posti di lavoro. Rischiamo un'ecatombe occupazionale ed è necessario intervenire con misure strutturali; cosa che questo e i precedenti decreti-legge non hanno mai fatto. Dobbiamo dire qualcosa anche sull'articolo 28, il caso del superbonus, indice di come opera questo Governo. Tutti siamo stati d'accordo nel dire che le truffe vanno frenate, frenate, evitate, ma evidentemente, se ci sono state, c'è un solo responsabile: questo Governo, il Governo dei migliori. Peraltro, l'Agenzia delle entrate ha parlato in modo chiaro

per cui l'accanimento che ha portato a circa 14 modifiche in due anni per questo incentivo appare avere basi piuttosto fragili. L'auspicio è che i nuovi correttivi appena inseriti siano gli ultimi correttivi per dare alle famiglie e alle imprese italiane, che vogliono usufruire di questo incentivo, almeno la certezza del diritto, come dovrebbe accadere in uno Stato civile. Purtroppo, con questi interventi fatti in nome del contrasto alle frodi, il Governo è riuscito a colpire uno dei pochi settori che mostrava un autentico rimbalzo, quello dell'edilizia. Se nel 2021 il PIL è aumentato del 6,5 per cento, ciò è dovuto per un terzo al settore delle costruzioni, che hanno segnato nel solo anno passato un aumento della produzione del 24 per cento, dell'11,8 dell'occupazione, del 27,7 delle ore lavorate e del 16,4 degli investimenti. in maggiori introiti per le casse dello Stato, così come hanno certificato anche gli Uffici del bilancio, per quanto riguarda IVA, Irpef, Ires e IRAP. L'articolo 28 chiaramente è stato superato dalle disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 13 del 2022. Infine, il tema della rottamazione-*ter* e del saldo e stralcio: è vero, c'è stato

quindi, serve andare oltre, serve più coraggio. Non basta la misura del differimento di un termine, tra l'altro di pochi mesi.

convinto che la rottamazione-*quater* non si possa fare perché non ci sono le risorse. L'auspicio è che la tendenza si possa finalmente invertire, senza attendere ulteriormente la fine delle emergenze che interessano il pianeta, anche perché, oltre all'emergenza pandemia e a quella legata alla guerra, rischiamo di aggiungere un'emergenza democratica: un'eventualità che tutti vorremmo e dovremmo scongiurare.

vorrei cominciare da una nota positiva, perché penso sia giusto e doveroso farlo. Mi riferisco al fatto che, sia pure con una distanza di tre mesi dalla legge di bilancio 2022, approvata alla fine di dicembre, il Governo ha finalmente inteso dare seguito all'impegno che aveva preso con Fratelli d'Italia quando, nel

che finalmente dà una risposta ad oltre 500.000 italiani onesti, ai quali si era chiesto di pagare, in un mese e mezzo, quello che non avevano potuto evidentemente pagare in quasi due anni di *lockdown*. Dispiace, però, dover dire che, nonostante l'emendamento fosse di Fratelli d'Italia, nonostante l'ordine del giorno originario fosse di Fratelli d'Italia, il primo partito presente in questo Parlamento, il MoVimento 5 Stelle, abbia tentato di appropriarsi anche di questo sul principale giornale nazionale. È davvero una caduta di stile, che non dovrebbe

E ribadisco che un partito, per di più il primo partito presente in Parlamento, se n'è appropriato sul primo giornale economico nazionale. Veramente dispiace. Dispiace perché l'etica e la correttezza, pur nel confronto politico anche più aspro, dovrebbero appartenere a ciascuno di noi. Quindi, una nota positiva, che però viene coperta da un atto di scorrettezza che non abbiamo gradito. Ci dispiace, lo ribadisco e lo sottolineo. Detto questo, entriamo nel merito delle vere problematiche. Il collega Calandrini, Capogruppo di Fratelli d'Italia in Commissione bilancio, è stato abbastanza chiaro nel denunciare, di fatto, come questo decreto di sostegno abbia solamente il nome, ma non certo i fatti: o comunque i fatti sono ben pochi. Ci troviamo, infatti, nel bel mezzo di una tempesta finanziaria, dovuta all'articolo 27, al problema dei crediti d'imposta. Il Governo già ha mille problemi da risolvere, lo comprendiamo: problemi legati alla pandemia, alla crisi politico-energetica, alla crisi internazionale che ha aggravato tutte le altre crisi. Ebbene, in tutto questo marasma, il Governo ha trovato modo di mettere in crisi un percorso, quello dei *bonus* edilizi, che era virtuoso, che tutti noi ritenevamo virtuoso. Lo ha fatto in modo inconcepibile e assurdo. davvero inconcepibile e assurdo. Anche le misure di correzione, individuate poi nel cosiddetto decreto bollette, non sono servite di fatto quasi a nulla. Sono abituato a parlare anche per dati di fatto. Mi giungono, in

Banca Popolare di Sondrio, ITAS Assicurazioni, primario *competitor* assicurativo italiano, Mediocredito, Banca di credito cooperativo di Verona e Vicenza, casse rurali e le altre banche nazionali, Unicredit e Gruppo Intesa sono in via di esaurimento. Questo è il dato di fatto che testimonia il vostro fallimento. Avete sbagliato. Nel decreto-legge sostegni avete fatto un danno irreparabile al sistema e nel decreto-legge bollette non siete neanche stati capaci di ravvedervi e di rimettere in pista in modo corretto il percorso che caratterizzava i *bonus* e i superbonus Quel che è peggio è che chi ci rimette in tutto questo è il Paese intero. Sono le imprese italiane: le imprese di costruzioni, le imprese legate all'edilizia, le società finanziarie che avevano lavorato nella cessione dei crediti, i cittadini, che trovano i cantieri bloccati, che non riescono ad andare avanti e che, nella migliore delle ipotesi, oggi, grazie ai vostri provvedimenti, signor Sottosegretario, si trovano di fatto a dover svendere il credito e, quindi, a prendere molto meno di quello che lo Stato investe. Altro che 110 per cento! Stiamo andando verso percentuali del 60-70 per cento quando va bene, perché nella maggior parte dei casi oggi non riescono più nemmeno a portare a casa un euro.

caso era prevista una norma semplicissima che di fatto ha retto. Mi riferisco al visto di conformità: professionisti *ope legis* obbligati all'assicurazione che, controfirmando una pratica, ne garantivano l'esistenza; infatti,

dove non era presente nemmeno un controllo. Serve il Governo dei migliori per prevedere che, se c'è un'agevolazione di peso, se ci sono crediti d'imposta dello Stato, un minimo di controllo deve esserci?

Dovevate semplicemente capire che il credito va identificato all'origine, va tracciato su una piattaforma finanziaria nei suoi passaggi e va corredato del visto di conformità. Con i passaggi identificabilità, provenienza (particella X e Y), tracciabilità del percorso di cessione (che quindi può essere infinito, se viene mosso sulla piattaforma finanziaria) e visto di conformità il Governo di sarebbe tutelato, avrebbe tutelato l'Erario, avrebbe tutelato i cittadini e avrebbe evitato gli sprechi. Invece, nonostante Fratelli d'Italia, con la sua opposizione costruttiva, lo abbia sempre detto, avete deciso di limitare la cessione dei crediti, che non serve a nulla se non a distruggere una misura. pertanto alle forze politiche che sono al Governo, che siedono in questo Parlamento e che sono convinto la pensino come me su questo. Non basta che lo dicano come facciamo noi, perché noi non abbiamo altro mezzo che poter parlare, salvo poi qualche volta venire espropriati anche del nostro lavoro. Voi siete al Governo, voi avete il dovere di cambiare queste cose! Avete il dovere di porre fine alla

per riprendere anche le parole del collega Calandrini e tanti ragionamenti svolti anche da altre forze politiche, il presente decreto-legge sostegni

Su questi temi vorremmo si misurasse il Governo; su questi temi saremmo felici che il Governo venisse etichettato come Governo dei migliori; ne saremmo felici noi dell'opposizione perché vorrebbe dire che in quel caso il nostro Paese e i nostri concittadini avrebbero le risposte che meritano, ma ahimè purtroppo oggi non è così.

circa un secolo fa Mahatma Gandhi ci ricordava la necessità di non aspettare che finisse di piovere, ma di imparare a danzare sotto la pioggia. Io credo che la stagione che abbiamo alle spalle e nella quale siamo immersi in questo momento sia una certificazione plastica di questa necessità. Dopo due anni di situazione drammatica, nel corso della quale il nostro Paese, insieme a tutto il mondo, potremmo dire, si è trovato a dover fronteggiare le ricadute e le ripercussioni di una pandemia che ha segnato in modo devastante il decorso della vita delle persone, siamo qui a convertire il

ciò che sta accadendo in Ucraina ha creato ripercussioni pesantissime sull'economia globale e soprattutto su taluni aspetti della vita. Il provvedimento mette in campo risorse che sarebbero importanti, ma che, a fronte

connessi al costo dell'energia e del gas, ma finalizzate ad aiutare anche molti settori che hanno vissuto e stanno vivendo una situazione davvero complessa: dal settore dell'Horeca, al settore del tessile e della moda, del turismo, della cultura, dello spettacolo, dello sport; gli enti locali, tutto il segmento della salute, le istituzioni sul territorio e il settore del trasporto. Di fronte al quadro di complessità che ci si trova a dover affrontare, è evidente che le risorse che il provvedimento prevede sono sono insufficienti. Chi ha lavorato nei giorni scorsi al decreto-legge si è reso conto che nei fatti, al di là di alcuni accordi complessivi da parte della Commissione, si è lavorato sul piano normativo per risolvere problemi, per togliere impedimenti e limitazioni, dando sostegno e agevolazione a determinati settori.

complessità della crisi energetica acuitasi a seguito delle vicende belliche che tutti conosciamo. Tutto questo anche per ottenere a livello europeo le autorizzazioni alla proroga per il *temporary* *framework*, affrontare il tema dell'autotrasporto, del sostegno ai del sostegno ai familiari delle vittime legate ad impegni connessi al Covid, tutto il lavoro di sostegno assolutamente necessario e fondamentale agli enti territoriali, al settore del turismo e della scuola. il comparto agricolo, il provvedimento prevedeva un intervento sul settore suinicolo, che pareva essere in quel momento il settore più in crisi. È evidente che ciò che sta accadendo in queste settimane con l'esplosione, da una parte, dei costi dell'energia e, d'altra, di tutti di tutti i costi connessi alle materie prime (dai fertilizzanti ad operazioni molto semplici, quale potrebbe essere l'irrigazione, che con i costi del carburante agricolo che stiamo vedendo in queste ore diventa una pratica praticamente insostenibile) richiedono e richiederanno un intervento fortissimo. Credo che la previsione di questo ordine del giorno e

tante, troppe sono ancora le domande che aspettano risposta. Se guardiamo complessivamente la strategia che prevede il provvedimento alla Camera sulle questioni energetiche, i provvedimenti in preparazione da parte del Governo e il provvedimento prossimo che dovrà essere emanato sulle questioni agricole, penso che cominciamo a intravedere una strategia complessiva, che poi scommetterà soprattutto sulla speranza che questa situazione di

tra cui vorrei anch'io ricordare le nuove possibilità per tutti i contribuenti italiani offerte dalla rottamazione-*ter*, saldo e stralcio. Con questo provvedimento, i termini per pagare le rate scadute si sono riaperti per tutto l'anno 2022. Vorrei porre l'attenzione su un emendamento approvato dalla Commissione e dal Governo che finalmente dà

senatori, gli aumenti dei prezzi nel settore dell'energia continuano e continuano con i conseguenti effetti negativi sulle imprese, oltre che sulle famiglie, naturalmente. Ecco perché, mi permetto di insistere, come ormai faccio da settimane, sulla proroga della moratoria sui mutui pre-Covid. Siamo soddisfatti della condivisione unanime di tutta la maggioranza parlamentare che, nell'ordine del giorno a questo decreto, ha impegnato il Governo ad adoperarsi presso le istituzioni dell'Unione europea affinché il quadro temporaneo UE (*Temporary Framework*) venga esteso e potenziato anche al fine di consentire la proroga della moratoria in favore delle micro, piccole e medie imprese relativamente all'apertura di credito e concessione di prestiti e finanziamenti. di prestiti e finanziamenti. Però questo non può restare un mero proclama e quindi vigileremo affinché il Governo, al primo decreto utile, in tempi brevissimi, approvi questa moratoria mutui per salvare migliaia migliaia di imprese dal fallimento. Questo è un risultato che premierebbe non tanto i partiti politici, ma le migliaia di imprese italiane che stanno soffrendo in questo momento a causa dell'insostenibile aumento dei costi, specie dell'energia, per la difficoltà nell'approvvigionamento delle materie prime o perché le loro attività sono praticamente ferme da dicembre, come è il caso del comparto turistico. Tale moratoria converrebbe anche allo Stato che, in assenza della quale, potrebbe ritrovarsi a dover fronteggiare una forte esposizione debitoria. Grazie alla precedente concessione, da parte del Governo, di sospensioni e dilazioni, il sistema bancario ha potuto beneficiare di un corposo intervento di garanzie statali.

che si siano avvalsi di tali garanzie statali e, conseguentemente, le banche creditrici sarebbero tenute ad attivare queste garanzie rilasciate in loro favore rendendosi così concreti gli oneri finanziari per i bilanci pubblici. Non esistono quindi profili di potenziali oneri a carico dei bilanci pubblici derivanti dalla proroga di misure di moratoria. Anzi, è vero il contrario, poiché senza una misura di questo tenore l'attivazione diffusa garanzie statali rilasciate determinerebbe immediati e difficilmente fronteggiabili oneri per i bilanci pubblici. Alla luce, quindi, del perdurare dello stato di crisi, acuito dalle tensioni registrate sul fronte dei costi delle materie prime e dell'energia, come appena ricordato, diviene necessario adottare questa moratoria per prorogare il termine di sospensione dei rimborsi almeno fino al 31 dicembre di quest'anno con effetto retroattivo al 1 gennaio. Abbiamo il dovere di scongiurare la chiusura di migliaia di imprese che, schiacciate dal caro bollette, sono impossibilitate non solo a fare investimenti ma financo a far fronte alle normali spese correnti. Gli aiuti previsti, pur rappresentando uno sforzo apprezzabile del Governo, non sono ancora sufficienti a fronteggiare la crisi economica di liquidità che stanno attraversando molti comparti e soprattutto - perdonatemi se lo continuo a rimarcare - quello del turismo. Occorrono pertanto continuità

e che dobbiamo occuparci prioritariamente dei profughi e delle devastanti conseguenze sull'economia, ma mi preme farvi notare che anche qui da noi c'è già stata la guerra: una guerra epidemica dagli effetti che tutti conosciamo. E c'è chi, in questa guerra, ha combattuto per noi ed è caduto per regalarci la possibilità di ritornare alla normalità. Non voglio pensare che siano egoismi di bottega, perché è stato proposto dalla Lega, a far sì che non venga riconosciuto adesso, senza se e senza ma, alle famiglie dei medici deceduti nella prima fase del Covid un giusto ristoro. Per quanto ci riguarda, non è importante che si chiami emendamento Cantù

per le misure adottate e adottande per superare la carenza dei medici e per il conseguente abbattimento delle liste di attesa. Nessuno ne ha fatto una questione di primazia; l'importante è fare e fare bene. modo, per le nuove regole di ingaggio degli erogatori, compresi i medici di medicina generale, il cosiddetto DM 71 prevede una serie di importanti misure già proposte nel disegno di legge n. 2153 per il riordino dell'emergenza-urgenza preospedaliera ed ospedaliera del marzo dello scorso anno. Ben venga siano tenute in debito conto dal Ministero della salute le elaborazioni della Lega per il rafforzamento delle cure territoriali, a loro volta integrate con la continuità assistenziale che abbiamo già proposto nei nostri Così per il ristoro alle famiglie dei medici deceduti, purché sia approvato ora,

Dimostrate seduta stante che non è vero, recependolo, vista la preannunciata fiducia, nell'emendamento integralmente sostitutivo del provvedimento in discussione. Non abbiamo bisogno della coccarda, ma pensavamo che neppure il Governo ne avesse bisogno. Chiamatelo come volete, purché lo facciate, senza ulteriore differimento, perché proprio un anno fa abbiamo convenuto che si istituiva la giornata della memoria e che il Governo si sarebbe impegnato a reperire i fondi necessari per onorarli dignitosamente oltre a prevedere misure anche a favore delle restanti categorie di operatori sanitari e socio-sanitari direttamente coinvolti e per coloro che hanno subito importanti menomazioni permanenti all'integrità psicofisica non soggette a tutela. Tutto questo finalizzando le risorse necessarie correttamente e congruamente, posto che, come noi abbiamo avuto modo di rimarcare in ogni sede, tali non possono considerarsi quelle ad oggi stanziate dal Governo, con il pur apprezzabile primo passo fatto all'articolo 31 del decreto-legge n. 17 del 2022. Non vorrei che, per riconoscere la misura, si creasse una sovrastruttura che potrebbe assorbire parte di quanto stanziato, che già è insufficiente di suo, per mantenere se stessa. È ciò che si fa che definisce ciò che si è; dimostriamo che si fa e - scusate se insisto - che facciamo bene.

Signor Presidente, colleghe e colleghi, il decreto sostegni-*ter* arriva in un altro periodo difficile per il nostro Paese, nel pieno della quarta ondata di Covid, e contiene diverse misure di sostegno alle attività e al nostro tessuto socio-economico. Tra queste sono previste anche delle norme in merito al nostro sistema sanitario. In particolare, si incrementa di 400 milioni di euro per il 2022 il fondo istituito dal decreto fiscale e finalizzato al ristoro di Regioni e Province autonome delle spese sanitarie collegate all'emergenza Covid, che aveva una dotazione iniziale di 600 milioni di euro per il 2021. Interveniamo sugli indennizzi per gli effetti avversi da vaccino, estendendo, in conformità a quanto disposto da numerose pronunce della Corte costituzionale, l'indennizzo a coloro che, a causa della vaccinazione (anche facoltativa) anti-Covid, abbiano riportato lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psicofisica. Ci sono inoltre norme in materia di fascicolo sanitario elettronico e governo della sanità digitale; speriamo che sia la volta buona di vederli finalmente realizzati ovunque. l'accesso gratuito per gli alunni della scuola primaria ai *test* antigenici rapidi, oltre che nelle aziende sanitarie territoriali, anche in farmacia o in strutture convenzionate (norma finanziata con uno stanziamento di ulteriori 19 milioni di euro). Ma non voglio parlare ulteriormente di quanto c'è all'interno di questo decreto-legge; preferisco parlare piuttosto di quello che manca. Manca una norma relativa all'assistenza sanitaria integrata, le cosiddette polizze di *welfare* aziendale, volte a rendere nulle quelle clausole che obbligano il cittadino a rivolgersi esclusivamente ai centri convenzionati per l'erogazione delle prestazioni. Il parere del Ministero dello sviluppo economico desta però non poche perplessità per la bocciatura dell'emendamento - aggiunge l'articolo 21-*bis*, con il quale viene prevista la nullità di «qualunque pattuizione o clausola che, nei contratti di assicurazione sanitaria a beneficio del lavoratore stipulati fra datori di lavoro e imprese assicuratrici, obbliga i lavoratori ad avvalersi di professionisti e strutture convenzionate con le imprese assicuratrici. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. Le previsioni contenute nelle clausole nulle sono sostituite di diritto da previsioni che consentono al lavoratore assicurato di avvalersi delle prestazioni di un professionista o una struttura non convenzionati con le imprese assicuratrici e di ricevere il rimborso del corrispettivo pagato o di parte di questo. Il rimborso del corrispettivo pagato dal lavoratore a favore di un professionista o struttura non convenzionati non può essere inferiore a quello previsto dall'impresa assicuratrice per il medesimo tipo di prestazione in caso di tutela assicurativa diretta, fermi restando i massimali e i limiti contrattualmente previsti. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai nuovi contratti (...)», eccetera. continua: nel merito, sentito il mercato assicurativo - lo sottolineo - si segnala il potenziale impatto negativo sulla libertà contrattuale delle parti e per i relativi effetti sui premi di polizza sui consumatori (ma la polizza la sottoscrive il datore di lavoro). In particolare, la previsione contrattuale di cui si propone la nullità ha funzione calmierante dei prezzi, consentendo di accedere alle offerte economicamente più sostenibili per i sottoscrittori. La medesima previsione contrattuale favorirebbe altresì l'ampliamento delle coperture assicurative - ma abbiamo detto che restava fermo tutto a quanto già previsto - con un'estesa mutualità del rischio e conseguente supporto al sistema sanitario nazionale (come se il supporto al sistema sanitario nazionale fosse qualcosa di negativo, invece che positivo). Il Ministero dello sviluppo economico, insomma, sembrerebbe aver formulato questo parere sentendo solo la campana delle assicurazioni: nessun cenno alle associazioni di consumatori o all'ordine dei medici, agli odontoiatri o alle sigle sindacali, trattandosi di polizze aziendali. Non va dimenticato poi che la calmierazione dei prezzi va solo a vantaggio degli introiti delle compagnie assicurative, che in questo modo si trovano a pagare di meno, perché ci sono meno prestazioni da rimborsare e non va sicuramente a vantaggio neanche dei centri odontoiatrici, per esempio, che erogano queste prestazioni, perché per fare i prezzi più bassi alle compagnie assicuratrici potrebbero essere costretti a utilizzare materiali più scadenti e manodopera meno qualificata, tutto a svantaggio del cittadino, che, quando ha un danno alla carrozzeria del proprio veicolo, può rivolgersi al carrozziere di propria fiducia, mentre, quando si tratta di farsi mettere le mani in bocca per farsi curare i denti o sul proprio corpo per altre prestazioni sanitarie, deve rivolgersi esclusivamente ai centri convenzionati. Mi avvio a concludere, Presidente: peccato che clausole di questo tipo siano già state giudicate vessatorie per ben due volte nel 2017 dal tribunale di Torino per quanto riguarda le RC auto; non si capisce come mai dovrebbe essere diverso il concetto quando si tratta di tutela della salute. *(Applausi)*. Solitamente cerco di essere pacata e *politically correct* nei miei interventi, ma di fronte a tanta spudorata faziosità - scusatemi - mi indigno profondamente e credo che ve ne siate accorti. Ho già ripresentato l'emendamento al disegno di legge concorrenza, perché la tutela della salute dei cittadini viene prima di tutto e non mi fermerò finché non lo capirà e accetterà anche il Ministero dello sviluppo economico. Invito tutti i colleghi che siano interessati all'argomento a supportare questa battaglia e a sottoscrivere il mio emendamento o a presentarne altri uguali. ringrazio, senatrice Pirro. I suoi toni sono stati vibranti e, nel contempo, le argomentazioni e le parole contenute,

i drammatici avvenimenti di queste ultime tre settimane hanno stravolto le prospettive precedenti e, di conseguenza, sconvolto le agende dei Governi dei Paesi europei e non solo, accelerando in maniera esponenziale i cambiamenti della situazione economica. Le dinamiche che tutti purtroppo conosciamo (i rincari dell'energia, del carburante e delle materie prime) comportano un aumento dell'inflazione molto preoccupante, attestata al 4,3 per cento, secondo i dati Istat di febbraio 2022 - lo ricordo - che però non tengono conto degli ultimi sviluppi. La situazione che stiamo vivendo implica che il Governo e il Parlamento debbano agire cambiando con rapidità le progettualità già previste e derivate dal quadro economico favorevole della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanze di novembre, chiuso a fine anno addirittura con un rimbalzo del PIL, sopra ogni aspettativa, al 6,3 Allora non c'era nemmeno l'ombra della scure della guerra e la campagna di vaccinazione faceva ben presagire per un'uscita dallo stato di emergenza. Determinante sarà quindi esaminare il DEF, con la fotografia aggiornata della situazione economica del Paese, rispetto anche al contesto internazionale, in tempi rapidissimi, per agire rispetto alle conseguenze non solo della pandemia, per cui questo provvedimento era stato concepito, ma anche della guerra. Ricordo che questa maggioranza si è coalizzata con l'unico obiettivo di uscire dall'emergenza da Covid-19 e per far decollare il PNRR; ora si trova ad affrontare quella che il presidente Draghi ha definito «un'economia di guerra». La nostra attenzione si deve concentrare prevalentemente su interventi per limitare l'inflazione, quindi a sostegno dell'impresa, per permettere una buona offerta, e dei cittadini, per dar loro più potere d'acquisto. sostegni-*ter* sono stati messi a disposizione 2 miliardi di euro, con cui essenzialmente si è provveduto a dare ulteriori sostegni ai settori particolarmente penalizzati dalla pandemia, stanziando risorse per ridurre i costi dell'energia per le imprese, ma oggi - è evidente - non basta più. buoni interventi, declinati in una serie di misure anche a vantaggio degli enti locali, ma devo evidenziare una criticità del provvedimento: l'intervento sul superbonus. Bloccando inizialmente le cessioni del credito, di fatto, si è bloccato tutto e non solo a partire dall'approvazione in Consiglio dei ministri del decreto-legge, ma fin dal suo annuncio. Questa è l'ennesima riprova che gli annunci anticipano gli eventi e le loro conseguenze. Tutto ciò, infatti, ha creato un terremoto, che ha colpito cittadini, imprese, istituti finanziari e tutto il complesso mondo coinvolto nella misura delle agevolazioni fiscali. Pur comprendendo la volontà del Governo di bloccare le frodi che sono avvenute grazie a queste agevolazioni (ricordo i circa 4 maggiormente imputabili al *bonus* facciate), non è possibile però bloccare una misura con effetti retroattivi, che ricadono anche su interventi già avviati, mettendo in seria difficoltà tutti, dal cittadino, che si vede costretto a pagare i lavori già concordati, all'impresa, che non può cedere il credito agli istituti finanziari. È vero che poi il decreto-legge è stato modificato, prevedendo ulteriori due cessioni del credito, ma è altrettanto vero che nel frattempo il sistema si è fermato per almeno due mesi. Ora, visto il momento che siamo costretti ad attraversare, credo sia importante sostenere le imprese e quindi il lavoro. Penso sia fondamentale, visti i rallentamenti subiti, prorogare subito la scadenza del 30 giugno, per dare certezze, che sono la base di una seria programmazione. Forza Italia ha portato importanti contenuti per migliorare il decreto-legge. Penso ad esempio - è già stato ricordato, ma è importante - alle remissioni degli inadempienti per problemi economici e alla rateizzazione della rottamazione-*ter*, a saldo e stralcio, con le dovute proroghe. evidente infatti che non si tratta di volontà, ma di impossibilità oggettiva di versare le tasse a causa della pandemia. Anche in questo modo si tutela chi lavora e crea lavoro e si consente la sopravvivenza di attività che altrimenti sarebbero destinate a morire. Signor Presidente, tengo anche a dire che dobbiamo davvero garantire il lavoro in questo momento. Per questo sarebbe stato opportuno approvare un emendamento presentato non solo da Forza Italia, ma anche condiviso ampiamente a un tavolo della maggioranza, alla presenza delle parti sindacali, che avrebbe permesso di continuare la somministrazione a tempo indeterminato per 100.000 lavoratori. Meglio garantire il lavoro a tempo indeterminato, anche se in somministrazione, o rischiare di lasciare a casa 100.000 lavoratori? È questo il rischio ampiamente denunciato, se non si interviene subito. A proposito di lavoro, consentitemi di ricordare, a nome del Gruppo Forza Italia e della nostra capogruppo Anna Maria Bernini, che fra tre giorni ricorrerà l'anniversario della morte di Marco Biagi. Vent'anni sono passati dalla sua tragica scomparsa, ma è impossibile dimenticare la sua visione del lavoro e di quella cultura del lavoro tanto attuale, che ancora e soprattutto oggi rimane fonte di ispirazione. Signor Presidente, Governo, colleghi, Il provvedimento su cui stiamo discutendo oggi è datato 27 gennaio e nasce per dare una risposta alle attività maggiormente colpite dalla pandemia, per dare ristoro a quelle che sono state chiuse, per contenere la diffusione del Covid e gli effetti diretti e indiretti dell'aumento dei prezzi, soprattutto quelli riferiti alle principali fonti energetiche. Il decreto-legge è stato pubblicato a gennaio, come dicevo, già in ritardo rispetto alle misure di contenimento di dicembre. Dal mio punto di vista, avrebbero dovuto essere contestuali, come ho già ribadito in un intervento precedente: quando

si sperava - che questa fosse la coda della pandemia e che, con l'arrivo della bella stagione, avremmo visto finalmente il ritorno a una pseudo-normalità, quindi il provvedimento in esame in questo momento è superato dall'ulteriore emergenza dovuta al conflitto in Ucraina, che ha decisamente peggiorato la situazione. le incertezze dell'andamento dei prezzi e la crisi di approvvigionamento delle materie prime ci impongono serie valutazioni, ma soprattutto azioni importanti per calmierare l'aumento del costo dell'energia e del gas, che impatta su famiglie e imprese, nonché sull'intera filiera dell'approvvigionamento. Il costo delle materie prime e l'aumento dell'inflazione mettono a rischio la ripresa del Paese, se non la fermano

Altre aziende stanno valutando questa ipotesi ed è evidente che non possiamo permettercelo. Se l'economia si ferma, rischia di morire,

ed è evidente che serve una forte iniezione di liquidità. I decreti che vengono emanati in questo periodo di ulteriore emergenza trovano le risorse all'interno del bilancio, che, com'è facile comprendere, non sono inesauribili ed è evidente come sia necessario ipotizzare un suo ulteriore scostamento; valutare insieme insieme all'Europa di mettere in campo anche nuovi strumenti, come l'eurobond; adoperarsi presso le istituzioni europee affinché il quadro temporaneo

le aiutiamo prorogando queste moratorie, non ce la faranno da sole, quindi ci dev'essere un impegno da parte del Governo per raggiungere quest'obiettivo. Calmierare e contenere gli aumenti di gas ed energia devono essere le azioni prioritarie di questi mesi, perché non solo produrre, ma anche trasportare le merci con questi costi non è sostenibile. Famiglie, imprese ed enti locali, con relativi servizi, sono già in difficoltà e non possiamo fare affidamento sulla loro resilienza, perché questa è già stata provata dalla pandemia. Forte è la preoccupazione e l'allarme viene anche dal mondo dell'agricoltura; per l'approvvigionamento di concimi e mangimi e per l'aumento dei costi dell'energia e della benzina e del gasolio (che serve anche per il trasporto). devono varare misure urgenti, perché questo serve a garantire la sopravvivenza dei prodotti *made in Italy*. È un comparto vitale, che, oltre all'aumento dei costi, deve affrontare il problema della diminuzione di produzione per la siccità. Tornando al provvedimento sostegni-*ter*, possiamo esprimere soddisfazione per gli emendamenti che prima citava il relatore Misiani: l'esenzione

perché alle volte semplificare significa anche far risparmiare i cittadini, perché la burocrazia è un costo. Quindi, il nostro lavoro era volto a fare questo, perché le risorse a disposizione dei parlamentari erano poche e ne siamo tutti consapevoli; però sulla semplificazione bisognava dare risposte più attinenti

dell'efficientamento energetico e dell'approvvigionamento da fonti rinnovabili. Oggi vedo che tanti colleghi finalmente parlano di superbonus al 110 per cento riconoscendo il lavoro enorme fatto dal MoVimento 5 Stelle su questo straordinario provvedimento.

sembra proprio la sagra dell'ipocrisia, lo voglio dire con chiarezza: davanti a un conflitto che scoppia in prossimità del confine del Paese, e nessuno se l'aspettava, con il Covid che ci ha già piegato in due dal punto di vista sanitario, sociale ed economico, evidentemente i sostegni diretti a imprese, famiglie e cittadini andavano dati con un decreto-legge cosiddetto sostegni; ma se tutti quanti continuiamo a parlare di efficientamento energetico, di fonti rinnovabili e poi, alla prima occasione, non facciamo su questo tema, siamo veramente ipocriti. *(Applausi)*. Attenzione, non mi riferisco a questo consesso, perché almeno ci ragioniamo; in Commissione ci confrontiamo, abbiamo preparato tutta una serie di emendamenti e alcuni li ricorderò. Quella che voglio ricordare oggi è la posizione del Governo qui rappresentato dalla Sottosegretaria. Stamattina il ministro Cingolani ci ha detto che resta valido l'impegno della riduzione entro il 2030 del 55 per cento delle emissioni, ma cinque giorni fa precisava: «Questo momento storico ci fa rendere conto di quanto sia importante ridurre gli sprechi. Il risparmio energetico è un comportamento intelligente, rispettoso di chi è meno fortunato di noi e un pilastro della transizione ecologica». Lo stesso presidente del Consiglio Draghi, con l'informativa alle Camere del 25 febbraio scorso, davanti alla crisi del gas, nel lungo periodo sta nel procedere spediti, come stiamo facendo, nella direzione di un maggiore sviluppo delle fonti rinnovabili». Il 9 marzo si soffermava sulla crisi energetica e sulla transizione ecologica dicendo: «essenzialmente la risposta è dare ora efficace e rapida diversificazione» e «sono stati messi in campo significativi incentivi per la sostituzione di impianti alimentati da impianti fossili a impianti rinnovabili, comprese le pompe di calore». Incentivi a pompe di calore, riduzione degli sprechi, risparmio energetico, maggiore sviluppo delle fonti rinnovabili e diversificazione delle forniture: tutte parole, bellissime parole. Per fare una transizione ecologica, però, innanzitutto realizzare una vera transizione energetica del Paese, che si può fare soltanto se avviene in ogni comunità. Per fare questo, è necessario che la transizione investa in maniera attiva e partecipe ogni cittadino,

una semplicità unica. Avremmo dovuto potenziare quegli strumenti nella conversione di questo decreto-legge e invece il Governo non ce li ha fatti potenziare. È vero, la colpa non è di questo o di quel partito: è del costo, ma i cittadini lo devono sapere. Come ci abbiamo provato? Noi abbiamo posto sul tavolo una serie di emendamenti, condivisi anche trasversalmente dalle forze politiche: il primo obiettivo tra tutti era cercare di eliminare il blocco della cessione dei crediti da parte di Poste e

ripristinare il principio della circolazione illimitata dei crediti, poiché, dopo il primo passaggio, sono diventati certificati e quindi certi. Vi è poi la questione della revisione del regime sanzionatorio per i tecnici asseveratori, i quali soffrono.

ricordare, innanzitutto, che su queste battaglie il MoVimento 5 Stelle per troppo tempo è rimasto solo. Ben venga l'aiuto di tutti noi a portare avanti queste iniziative. Stamane, però, il ministro Cingolani nella sua informativa ci ha ricordato una serie di punti. In particolare, ci ha parlato della diversificazione delle fonti energetiche

dal colpire gli extra profitti dei produttori di carburanti, che in questo momento stanno toccando cifre a tantissimi zeri. Noi chiediamo di fare un fondo *ad hoc* per imprese, famiglie e autotrasportatori. Mi aspettavo dal ministro Cingolani che oggi ci parlasse anche del decreto ministeriale che ha firmato in data 14 febbraio 2022, relativo ai massimi prezzi per la congruità dei prezzi dei *bonus*. Perché non è stato ancora pubblicato, dopo oltre un mese, in *Gazzetta Ufficiale*?

la produzione da fonti rinnovabili nel nostro Paese, ci vedano uniti. All'unanimità dobbiamo far capire al Governo che quella è la priorità per la nostra politica.

è il disinteresse più totale alla trattazione del provvedimento da parte dei colleghi. È ovvio e naturale che, dopo 44 voti di fiducia, il parlamentare smetta di fare appello al senso di responsabilità, alla voglia di lavorare e di applicarsi, allo studio e all'elaborazione dei provvedimenti, al sostegno del dibattito prima in Commissione e poi in Aula. Smette di fare il suo lavoro e questo è

Chi? Chi ce li deve mettere questi soldi? Sono soldi spesi dalle Regioni, non promessi; sono spesi, già rendicontati. Chi più furbo, chi meno furbo, ma voi dovete controllare, siete deputati a questo. Chi più furbo, chi meno furbo, si tratta comunque di denaro rendicontato. Come fate a dire di mettere 400 milioni a titolo definitivo? Come a titolo definitivo? Allora le Regioni vanno in dissesto. Devono andare in dissesto. Voi state annunciando che tutte le Regioni d'Italia andranno in dissesto.

Non c'è più trippa per gatti. Da dove viene quest'arroganza nei rapporti istituzionali? Dov'è la sana e corretta collaborazione tra le Istituzioni e gli enti? Dov'è? E come mai si è così sicuri che si può parlare in questo sciagurato Paese a titolo definitivo? Qui di definitivo non c'è niente. Ci sono solo la vostra incapacità e la vostra inconsistenza, senza alcuna

Riconoscete che si devono indennizzare gli eventi avversi da vaccini per chi si è vaccinato fuori dall'obbligo (che, presupponendo un trattamento sanitario, è quindi già indennizzato di suo, forse). Mettete quindi denaro per indennizzare gli eventi avversi da vaccini. Bene, sapete quanto date per l'evento avverso ai familiari

diciamo per colpa dell'epidemia, se vogliamo l'attenuante generica. Ancora stiamo a litigare sugli indennizzi dei sanitari deceduti a causa della prima e della seconda ondata del Covid.

Avete deciso di finanziare le mascherine per gli studenti, senza chiarire che è lo Stato che deve fornirle. Le avete

di lamentele e rampogne, è giusto anche che si chiuda con un moto di speranza, almeno uno, che un emendamento approvato, proposto dal sottoscritto e da Fratelli d'Italia, che mette a disposizione una certa cifra in partenza per le famiglie e i soggetti costretti a usare attrezzature tecnico-medico-sanitarie,

è ancora peggio, perché significa che qualche volta, quando capite, le proposte serie sapete anche affrontarle. Allora fatelo sempre, Allora fatelo sempre, perché attraverso l'attività parlamentare - quella normale, non questa - i provvedimenti si possono solo migliorare e l'Italia può solo andar meglio, se le istituzioni funzionano.

del Parlamento, che in questo momento lei rappresenta, devo comunque dire che il Governo oggi è presente, attento e prende nota. Senza nulla Senza nulla togliere al suo diritto di dissentire, lo ribadisco, questo è proprio uno di quei casi in cui il Governo è assolutamente presente, attento e partecipe.

che sarebbe capitato e quello che stiamo vivendo oggi. Pensavamo ottimisticamente, anche con questo ulteriore decreto-legge che stiamo convertendo in legge, di poter dare ulteriore conforto e sostegno e sanare le tante problematiche economiche che si sono create a causa della pandemia. Mai avremmo pensato

dicembre 2022. Fino al 2021 era stata garantita la possibilità per i privati proprietari di immobili resi inagibili dal terremoto di non versare l'imposta municipale. Questo mio emendamento, a prima firma di alcuni colleghi ma presentato anche dal PD, ha portato finalmente

gratuiti per gli studenti. Penso anche all'articolo 20 che ha finalmente istituito un fondo indennizzi per le menomazioni derivate da vaccinazioni Covid che - se ricordate - per tanto tempo avevamo perseguito anche nei precedenti provvedimenti, non meno nella legge di bilancio. Qui lo vediamo scritto e, quindi, anche su questo tema c'è stato un accoglimento da parte del Governo.

che a questo punto diventa anche riferimento importante per quanto riguarda tutti i dati che saranno contenuti nei fascicoli sanitari elettronici che finalmente le Regioni dovranno

specializzandi la possibilità di collaborare a questa importante azione. Purtroppo il lavoro per uscire da questa crisi sarà ancora lungo, lunghissimo, e la sottosegretaria Guerra sa quanto si sta lavorando. Ma, a differenza di quanto si poteva pensare, l'obiettivo più grande - secondo me - quello che ci deve guidare, è avere un mondo senza guerra, per condividere tutto fra i popoli, la pace. *(Applausi)*.

Secondo me, la peste suina è incontenibile; se si allargherà alle Province vicine, a quelle di Alessandria e di Genova - ho qualche notizia proveniente da quelle parti - saranno miliardi. Il Governo prepari miliardi in qualche modo, stampi moneta, perché

è un macigno che ci sta davanti, perché tutto quello che può essere stanziato (oppure la facoltà di usare i ribassi d'asta) e le somme a disposizione sono importi troppo piccoli rispetto a quello che sarebbe necessario quando c'è un incremento superiore all'8 per cento (anche del 15-20 per cento), soprattutto per certi fattori. Forse conviene spostare la validità dei contratti e delle opere e sospendere un po' per tranquillizzare i prezzi.

dal 1° giugno o dal 1° ottobre 2021 o in procinto di essere collocati in quiescenza entro il 30 giugno o il 31 dicembre 2022, possano chiedere di essere richiamati in servizio o continuare il servizio per un periodo di dodici mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione. scritto in un italiano comprensibile anche all'italiano medio; io sono fautore di leggi che non si prestino al contenzioso, scritte in maniera che possano essere capite e attuate. Il Ministero ha redatto un emendamento, che è stato approvato gioco forza dalla Commissione e che è un po' più complicato - ma forse la natura di queste cose è così - in cui si dice che,

La categoria dei segretari comunali e provinciali è molto importante per gli enti, perché essi garantiscono la legalità e sono a supporto delle amministrazioni. C'è una classe sia anagrafica, sia di concorso, che sta per andare in pensione o che vi è già andata, per cui c'è un vuoto assoluto. Conosco delle situazioni

emendamento suggerito dal Ministero dell'interno prevede che il corso-concorso duri quattro mesi e sia seguito da un tirocinio pratico di quattro mesi.

mi sembra che sia un di più, ma sta bene anche questo. In ogni caso, la questione dei segretari comunali è importantissima; proporrei delle soluzioni semplici, per garantire la continuità del servizio.

va spostata, anche per dare tranquillità al settore. La tranquillità è anche una questione di tranquillità dei prezzi, perché calma un po' la speculazione.

prima della cessione dei crediti, per la quale ho avuto rassicurazioni dalla sua collega Sartore in Commissione: il meccanismo a cura di Sogei è in moto, perché dal 1° maggio ci vuole il codice, altrimenti le pratiche si arenano.

con una scadenza certa che dia la possibilità di finire i lavori e provare a ragionare, se possibile, e sovvertire un po' il principio della Ragioneria dello Stato per cui la quota da finanziare sia pareggiata dai maggiori incassi che determinano maggiori investimenti, mentre vanno a finire nel calderone dello Stato e non sono contabilizzati con questa finalità. Da ultimo, spero che il maxiemendamento recepisca i 90 emendamenti approvati dalla Commissione. Sottolineo anch'io che per me la fiducia è una cosa seria, come diceva una pubblicità di anni fa. Bisogna quindi trovare, gradatamente, un altro metodo.

del provvedimento che ci accingiamo a votare. Sicuramente questa è una delle poche volte in cui ci è capitato un provvedimento che non ha risorse, come è stato ben detto dal relatore nella sua esposizione. Effettivamente, visti i diversi passaggi, ci è toccato cercare di legiferare

possa dare un frutto povero, acerbo, che non ha significato. Invece, secondo me, è quando non ci sono i soldi

nella tensione di produrre un emendamento senza supporto economico, che magari apre un ventaglio di possibilità e riesce a risolvere una serie di situazioni completamente bloccate. A questo provvedimento sinceramente non ho presentato neanche un emendamento, ma ho seguito emendamenti di altri colleghi. Mi sono impegnata perché mi piaceva, perché era un cerebrale. Nel suo modo di essere cerebrale, se molti di quegli emendamenti fossero stati presi in considerazione in modo ben preciso, sicuramente avrebbero sollevato avrebbero sollevato e aiutato tantissime situazioni ancora irrisolte. Faccio un esempio: la senatrice Cantù ha parlato della questione dei medici, ma il suo era

Non c'erano i soldi, ma bisognava sicuramente metterci la testa in maniera più approfondita. Faccio l'esempio di quello della collega Fregolent, che era già a posto e che non si sa per quale motivo, nonostante ci fossero i soldi e il via libera del Ministero, si è perso. Torno allora a ripetere una cosa che ho già detto altre volte. Noi siamo in uno stato di emergenza economica, di salute, finanziaria e sociale. Dovremmo essere anche noi in uno stato di emergenza e mollare

e cercare di sistemare tutte quelle situazioni in cui, se per noi due mesi non sono niente, per quelli fuori invece sono tanti. Concludo il mio intervento rivolgendomi al simpaticissimo collega Zaffini di Fratelli d'Italia, che ha sciorinato tutta una serie di situazioni molto negative su come noi non siamo

perché solo così ha significato quello che lei dice in relazione a ciò che il suo partito sostiene al di fuori e dentro quest'Aula. Quanto agli altri non posso dire diversamente, perché effettivamente un provvedimento così, che non ha supporto economico, ma che ha forza per dare fuori, avrebbe dovuto vedere l'Aula piena, il sostegno ai relatori e alla Commissione, che ha cercato in tutte le maniere di fare quello che poteva, perché quelli che... devono assolutamente comprendere che il nostro non è un lavoro da stipendiati di alto lusso:

Il decreto-legge è stato pubblicato a gennaio in una situazione oggettivamente differente rispetto a quella attuale e si pensava che potesse essere la coda dell'emergenza da Covid-19.

e alle sue conseguenze sull'economia mondiale, al caro energia, alle incertezze sull'andamento dei prezzi e alla crisi di approvvigionamento delle materie prime. Emerge quindi l'urgenza di interventi più decisi in alcuni ambiti come il settore primario, quello della distribuzione e settori energivori, e ciò nonostante si sia riusciti ad agire sulla rottamazione-*ter*, evitando che migliaia di contribuenti e imprese venissero strangolati dalla fiscalità che - chiariamo - deve aiutare i cittadini e non ostacolarli. Rispondo anche all'amico e collega De Bertoldi di Fratelli d'Italia, che ha sollevato una polemica che non interessa tanto i contribuenti sulla paternità l'emendamento.

Per quanto riguarda il Gruppo MoVimento 5 Stelle - come ben spiegato anche dal principale giornale economico - abbiamo iniziato a gennaio a indagare

L'effetto combinato di un aumento generale del costo dell'energia, delle difficoltà di approvvigionamento di materie prime e dell'inflazione ci fa rientrare in un'emergenza nel momento in cui stiamo uscendo auspicabilmente da un'altra. Chi più ne sta soffrendo sono le piccole e medie imprese nel settore degli autotrasporti, a cui urge dare una risposta immediata in questo momento. Il Governo, quindi, deve essere impegnato su questo. Rispetto a quanto detto dal ministro Cingolani questa mattina, vorrei sottolineare alcuni aspetti positivi. Innanzitutto, mi preme evidenziare l'importanza del passaggio sulla accisa mobile. Credere, infatti, che il problema energetico sia una questione isolata dalle altre componenti della società è sbagliato, la natura regressiva delle accise. È evidente che il termine «regressivo» è stato utilizzato con facilità anche dal nostro Presidente del Consiglio per misure come il *cashback*, anche innocue da questo punto di vista - se vogliamo - mentre non ho sentito il termine «regressiva» L'accisa è una delle imposte più antipatiche da questo punto di vista e deflagra quando andiamo incontro ad aumenti del costo del carburante come quello che stiamo vivendo in questi giorni e rischia di creare situazioni drammatiche per le nostre imprese.

Per questo, una rimodulazione della tassazione, anche in virtù del maggiore importo derivante dall'IVA, è di fondamentale importanza, non fosse altro che per una questione di giustizia sociale: non possono pagare la crisi solo i cittadini. altro elemento degno di nota è certamente lo sganciamento del prezzo del gas dal costo dell'elettricità e su questo bisogna essere chiari: le rinnovabili convengono.

da fonti rinnovabili, perché ormai siamo arrivati a un punto della storia - per fortuna - in cui l'energia rinnovabile costa meno dell'energia fossile, per una semplice questione di esternalità positiva, di effetti sull'ambiente e di effetti sui portafogli dei cittadini. Oggi è ancora più importante che questa misura venga presa in tempi brevissimi, fin da subito, per godere degli incentivi naturali verso le rinnovabili. Voglio anche ricordare, però, che per numero di installazioni fotovoltaiche siamo secondi in Europa, dietro la Germania, ma abbiamo meno della metà del suo installato (22 gigawatt l'Italia contro i 55 gigawatt della Germania). Questo è un enorme controsenso, dato che siamo a tutti gli effetti una potenza solare maggiore rispetto a tantissimi Paesi e, in questo caso, alla Germania. A livello di installazione *pro capite*, invece, siamo al decimo posto in Europa. La domanda, quindi, è per quale motivo si è così ostacolato il superbonus. Il Ministro ha parlato del pacchetto RePower EU, ma i pilastri di queste misure non sono il risparmio energetico, la diversificazione delle fonti energetiche, l'indipendenza che è stata citata. Quale altra fonte può passare se non dalle rinnovabili e non sono queste le ragioni fondamentali alla base del superbonus stesso? A me sinceramente sorprende il fastidio che si prova verso il rendere autonomi i singoli cittadini. In Europa ci stanno seguendo e hanno capito che una delle strade principali da percorrere è l'indipendenza dei singoli, e quindi l'autoproduzione e l'autosufficienza energetica. È evidente che non risolve il problema dell'approvvigionamento energetico, ma è sicuro che riduce la domanda di energia. E non c'è bisogno di essere economisti per sapere che, nell'incrocio tra domanda e offerta, quando si riduce la domanda si riduce il prezzo. È una banalità, ma è alla base dell'economia. I dati ENEA ci dimostrano quale sia stato il vero impatto del superbonus, al di là di tutte le narrazioni politiche di questi giorni. A gennaio gli interventi finanziati tramite il superbonus hanno consentito un risparmio di energia elettrica pari a oltre 3 milioni di megawatt: si tratta del fabbisogno energetico annuo di 1,1 milioni di famiglie. Un altro punto importante evidenziato dal Ministro - lo sottolineo - è la liberalizzazione delle installazioni da rinnovabili fino a 200 chilowatt: una misura che deve essere strutturalmente accompagnata da un aumento delle detrazioni sui pannelli fotovoltaici e sui sistemi di accumulo. I cittadini che spesso sono più intelligenti di chi li governa hanno capito da soli che in questo momento conviene rendersi più autonomi possibili rispetto ai soggetti che controllano l'energia. Il costo dell'energia è decisamente fuori scala: non è più giustificabile alcuna attesa, le valutazioni sono fuori tempo massimo e i cittadini non possono aspettare ancora. è indispensabile che il Governo intervenga contro i fenomeni speculativi per tutte quelle filiere in ginocchio; altrimenti il rischio concreto è che si fermi il nostro Paese. *(Applausi).*

i colleghi Calandrini, Zaffini e De Bertoldi hanno già detto quello che Fratelli d'Italia pensa del provvedimento in esame, ma mi sia consentito dire avendo ascoltato con attenzione anche gli interventi dei colleghi degli altri Gruppi di maggioranza - che il provvedimento non soddisfa nessuno. Il decreto-legge esame avrebbe dovuto trovare e dare altre risposte ai settori della vita della nostra Nazione, invece il Governo manca di coraggio. La verità vera è che, per mettere in campo le risorse necessarie per dare risposte reali ed efficaci, dovrebbero presupporre impegni economici di altra natura, o quantomeno scelte politiche che vadano nella direzione opposta rispetto a quella che il Governo ha scelto: un nuovo scostamento di bilancio. Lo diciamo con la credibilità di chi, pur essendo forza di opposizione, ha dimostrato di essere capace di votare questa necessità necessità in altri tempi e momenti della pandemia. Non vogliamo aiutare il Governo - non ci convince mai, dal primo momento - ma non ci tiriamo mai indietro quando dobbiamo aiutare l'Italia e gli italiani. Mi chiedo a cosa serva un'attività emendativa da parte della maggioranza, quando si è consapevoli - già dal principio - che non c'è possibilità di intervento, anche su questo provvedimento. Oltre 2.300 emendamenti certificano in partenza che siamo al cospetto di un decreto-legge assolutamente insufficiente.

e poco gli cambia se il provvedimento si chiami ristori o sostegni, perché non avete cambiato la filosofia di intervento. I minuti che mi restano li voglio dedicare ad una questione che, come partito, abbiamo cercato di segnalarvi, nell'importanza che assume, cercando di stare almeno sull'emergenza, se non è possibile stare su una visione complessiva e strategica, che manca. Tra quattordici oltre 55.000 persone, che hanno mandato avanti la scuola italiana, vedranno scadere il loro contratto. Mancano

Noi ci siamo battuti con un emendamento. Avevamo speranza che si potesse risolvere questa problematica, per fare in modo che la scuola italiana potesse andare avanti. Non ci sono le risorse, dopo che erano state date tante speranze e si era detto che anche altre forze politiche avevano presentato lo stesso emendamento. Noi diciamo al Governo che ci vogliamo ancora credere.

onesti intellettualmente. Faccio espresso riferimento alla questione che ha consentito, con un nostro emendamento, di dare uno scudo, civile, penale ed amministrativo ai dirigenti scolastici. Bisogna fare uno sforzo per prorogare questo personale a giugno del 2022. Non promettete ancora cose che non farete o soluzioni confuse, calciando la palla in avanti e dicendo loro che troverete le risorse nel DEF, per prorogare di un mese fino al 30 aprile...

anche a 1.000 chilometri di distanza. Invece di dissipare miliardi in improduttivo reddito di cittadinanza e sussidi, facciamo in modo che chi ha lavorato, chi lavora e chi vuole continuare a lavorare nell'interesse dello Stato abbia la propria risposta. il provvedimento cosiddetto sostegni-*ter* abbia visto l'approvazione di 90 emendamenti in Commissione. Credo sia questa la testimonianza più importante del lavoro che è stato fatto in Commissione. Ringraziamo i relatori anche per quello che hanno riferito all'Assemblea, pur nelle difficoltà. Di questi 90 emendamenti, noi siamo particolarmente felici dell'approvazione di uno all'articolo 21, dedicato al fascicolo sanitario elettronico. È stata approvata, a mia prima firma, una proposta che stabilisce che ogni prestazione sanitaria erogata da operatori pubblici, privati accreditati e privati autorizzati, sia inserita entro cinque giorni nel fascicolo sanitario elettronico. Io mi rivolgo anche ai cittadini e alle cittadine in quest'Aula. Questa è una vera rivoluzione ed è la costruzione della sanità di oggi e della sanità Il fascicolo sanitario elettronico è la nostra carta d'identità sanitaria, condivisa con i professionisti sanitari per garantire un servizio efficace ed efficiente. Ognuno di noi può seguire il proprio percorso di salute e avere un accesso ordinato e aggiornato. Naturalmente sul fascicolo sanitario elettronico non si parte da zero. Ci sono molte Regioni e, quindi, anche qui scontiamo le differenze regionali. Ci sono 21 fascicoli sanitari diversi, ma con questo articolo 21, in generale, si mettono davvero le basi della sanità digitale e soprattutto si opererà con un linguaggio comune dei dati. Qui consiste la vera rivoluzione. Con l'emissione dei dati anche da parte dei professionisti della salute che operano in ambito privatistico viene ulteriormente perfezionato e arricchito il profilo del paziente. Questo consentirà ai medici e a tutto il personale sanitario di avere in tempo reale un completo quadro clinico aggiornato, cioè la nostra storia sanitaria, con refertazioni di patologie, patologie, disfunzioni, terapie farmacologiche, interventi chirurgici pregressi, radioterapie, fisioterapie, tutto. In prospettiva credo che sia di grande valore il fatto che questa norma sia stata approvata all'interno del terzo decreto-legge sostegni, perché dopo l'epidemia abbiamo il dovere morale, civico sociale di mettere a posto la sanità. Cito alcune questioni di prospettiva: riuscire a evitare la frammentazione diagnostica e terapeutica; ridurre il peso derivante dalla mancata adesione ai piani terapeutici, soprattutto degli anziani; validare e implementare la prevenzione e quindi ridurre i fattori di rischio con stili di vita corretti; evitare ripetizioni di accertamenti recenti; controllo della spesa sanitaria; verifica e conoscenza costante di eventuali intolleranze e allergie ai farmaci, che saranno tutte riportate nel fascicolo sanitario elettronico; unicità del paziente rispetto ai presidi sanitari pubblici e privati; miglioramento delle competenze digitali fondamentali per la transizione sanitaria, nel panorama di una comunicazione digitale ad uso e consumo della cittadinanza, nell'ottica di una sempre più moderna e innovativa sanità digitalizzata; verifica continua, attraverso il fascicolo sanitario elettronico, della *compliance* terapeutica del paziente, monitorando parametri fondamentali, riconducendo di conseguenza anche i costi di cura del paziente, minimizzando i disagi dovuti agli spostamenti sul territorio e offrendo una qualità di vita e di cura nettamente migliori. Con questo allargamento dell'obbligo di inserimento e di aggiornamento del fascicolo sanitario elettronico potremmo, infine, dare un grande aiuto al telemonitoraggio a domicilio dei malati, che consentirebbe di ridurre giorni di degenza, con un risparmio di costi sanitari, aumentando anche il tasso di sopravvivenza.

ha bisogno di altro; infatti un ordine del giorno della maggioranza chiede di reperire ulteriori risorse per un ulteriore provvedimento che sia di maggiore attualità.

delle cessioni di credito che avevano messo un po' in difficoltà tutti gli operatori del settore dell'ecobonus. Abbiamo provato a dare certezza su tempi, metodi e modi. Non siamo riusciti invece, come dicevo in

Nel codice degli appalti, approvato la scorsa settimana, abbiamo messo qualcosa di più concreto, che però darà frutti tra un anno, un arco temporale troppo lungo. È evidente che sull'argomento bisognerà tornare e mi pare che sul tema ci sia convergenza di Governo, relatori e parlamentari.

oltre 80 emendamenti approvati. Sul punto tornerò nelle conclusioni. Abbiamo introdotto poi alcune misure importanti e significative. Mi attengo soprattutto alla materia di competenza

presieduta dal presidente Atelli, come d'altra parte la Commissione generale VIA-VAS. Devo dire che fin qui vi è una chiara inversione di marcia nei tempi in cui tali Commissioni danno i propri pareri; cosa che va sottolineata perché in tanti altri casi si trattava esattamente del collo dell'imbuto. Abbiamo introdotto misure che la rafforzano. Avevamo chiesto anche un rafforzamento ulteriore, ma ci torneremo in altri casi. Insieme a quasi tutti i Gruppi, abbiamo presentato ed approvato un emendamento sul trasporto pubblico locale, anche questo di grande importanza. Diamo cioè la possibilità di prorogare i contratti in essere fino al 2026, garantendo così un orizzonte temporale a società di gestione del trasporto pubblico locale, a condizione che esse investano in autofinanziamento delle proprie risorse che, sommandosi a quelle del PNRR, possano produrre un effetto moltiplicativo di grande importanza di qui al 2026. Un altro importante emendamento riguarda le misure a supporto di Anas e delle imprese ferroviarie, di Ferrovie dello Stato, sia verso le imprese che trasportano merci, ma anche incrementando alcuni stanziamenti a favore di Anas per tener conto del calo di entrate dovuto negli anni scorsi alla minore circolazione.

infine, ma non per ultimo, segnalo un emendamento in favore dei medici che lavorano sulle navi mercantili o crocieristiche. Concludo con quanto avevo accennato all'inizio: mi pare un ottimo segnale che anche in questo caso, come nel provvedimento approvato la scorsa settimana, ci sia un numero elevato di emendamenti approvati in Commissione. Questo, Presidente, colleghi e Governo, è il modo virtuoso di lavorare in Parlamento. Il Consiglio dei Ministri svolge il suo ruolo, noi abbiamo il compito di intervenire sugli atti, migliorandoli ovviamente senza snaturarli, ma dando il nostro contributo di idee, di intelligenza, di competenza e di lavoro.

qualche collega negli interventi che mi hanno preceduto si è posto questa domanda: dov'è il sostegno in questo decreto-legge? Il sostegno non c'è; c'è solo qualche boccata d'aria per qualche settore completamente in ginocchio. Qualche altro collega ha detto: abbiamo lavorato con il Governo. Ma chi ha lavorato con il Governo? Ancora una volta, anche in questo provvedimento, il Parlamento è stato completamente esautorato. Ciò che sta accadendo in queste settimane non lo ripeto; a livello geopolitico l'abbiamo detto e l'hanno ribadito un po' tutti. Però quello che sta succedendo in agricoltura, materia di competenza della mia Commissione, ci fa capire quante scelte sbagliate sono state fatte negli ultimi anni anche nella politica agricola, politica agricola, sia nazionale che europea, ed ora ne stiamo pagando le conseguenze. Siamo infatti in balia di una incontrollata speculazione messa in atto sui mercati, che, da un lato, ha portato all'aumento esponenziale dei prezzi e, dall'altro, ha portato ad una carenza senza precedenti nelle materie prime. Le piccole e medie imprese della pesca e dell'agricoltura non ce la fanno più; non ce la fanno assolutamente a far fronte alle spese per il costo del gasolio e per l'acquisto delle materie prime, fosse anche solo per organizzare la prossima campagna produttiva. In questo momento serve liquidità alle aziende. La liquidità alle piccole e medie aziende, sia agricole che ittiche, si sarebbe potuta assicurare con un emendamento da me presentato a questo provvedimento; da me presentato, ma fortemente chiesto da tante piccole e medie imprese disperate che si sono organizzate in un coordinamento nazionale spontaneo (Copoi) del quale sono referente. Questo emendamento all'articolo 3 - lo troviamo all'interno del fascicolo degli emendamenti segnalati - chiedeva non un *bonus* o un regalo, ma semplicemente un finanziamento della durata di dieci anni

C'è chi dice che non ci sono soldi, ma in una situazione del genere potremmo anche pensare a uno scostamento di bilancio.

ma poi questi stessi soggetti collaborano e si coordinano per destinare ingenti somme di denaro ad infrastrutture magiche, costruite ad arte e *ad hoc* in tutti questi anni, nei cui meandri si perde tutto: soldi, progetti e quant'altro. Tutto questo senza che agli agricoltori arrivi almeno il costo di produzione; nemmeno quello abbiamo garantito in questi anni, tant'è vero che determinate filiere sono state abbandonate - parlo della filiera del grano e del mais perché agli agricoltori non è stato assicurato il costo di produzione e adesso ci troviamo sotto scacco rispetto a tante situazioni e a tante filiere. Quindi ancora una volta ho dovuto dire al mondo delle piccole imprese agricole e dei pescatori, che hanno fermato i loro pescherecci perché non ce la fanno a garantirsi il gasolio, che non ci sono soldi. Naturalmente la risposta che mi danno è questa: cara senatrice, quando i soldi li vogliono far uscire per indirizzarli dove vogliono loro, i soldi ci sono ed escono.

di osservazione che magari non vanno nell'indirizzo di esprimere solo un plauso, visto che non siamo qui ad auto-applaudirci, ma a cercare di evidenziare le criticità. Evidentemente il decreto-legge in esame è nato in un tempo non sospetto, precedente alla guerra, e già di per sé

la risposta del Parlamento e del Governo sia molto lenta rispetto ai problemi che si vivono quotidianamente fuori da questo Palazzo. Immagino che ciascuno di noi vada sui territori e incontri le persone, le famiglie e le aziende.

sue dinamiche sono apparse risibili o distanti dalla realtà, quella vera e reale che c'è fuori da questo Palazzo. Dire di no semplicemente perché la relazione tecnica non è pervenuta è ridicolo e fuori dal mondo e vuol dire non capire quello che sta accadendo fuori di qui. Dire di no semplicemente perché non si è fatto in tempo a fare un'istruttoria è inaccettabile.

Questo deve essere chiaro a tutti quanti noi. Non siamo qui lo scendiletto di alcuno. Se non siamo in grado di difendere le battaglie che, da fuori, portiamo dentro il Palazzo e al Governo siamo del tutto inutili. Non è tollerabile che ci sia una relazione tecnica non pervenuta. Si dice che noi difendiamo le aziende. Quali aziende? Quelle con fatturato sopra i 50 milioni di euro? Quelle aziende non sono la spina dorsale del Paese. abbiamo presentato emendamenti per rafforzare il patrimonio delle medie imprese e più volte ci è stato detto che l'istruttoria non si è completata.

Chiedo al Governo e soprattutto al Parlamento di essere coerenti quando lanciamo i moniti, perché altrimenti rischiamo di fare la sceneggiata per cospargerci la testa di cenere.

Quante sono le aziende in Italia con fatturato sopra i 50 milioni? L'altro tema che ho posto in Commissione riguarda le strutture sanitarie. Tutti gli assessori regionali alla sanità hanno chiesto alle aziende private e pubbliche di costruire degli edifici per l'emergenza. Dopo tanti tagli

Che fine fanno queste strutture? Il primo funzionario dell'ufficio edile di un qualunque Comune che si alza e va a fare un'ispezione è costretto a chiedere l'immediata rimozione della struttura. Anche in questo caso non c'è stata la possibilità di intervenire per dare loro certezza e, come per tutte le cose belle che avvengono in questo Paese, bisogna sempre creare l'incertezza, perché nell'incertezza spunta fuori il provvedimento di emergenza. Forse talvolta potremmo prevenire

lavorare su un decreto-legge superato nei fatti dagli eventi. Ma in questi due anni c'è stata un'accelerazione di eventi che hanno sconvolto il normale andamento della vita delle famiglie, delle imprese, dello Stato e dei Comuni. Occorre quindi andare veloci e cercare di intervenire con provvedimenti puntuali e con una celerità volta proprio a evitare che il sistema salti. l'inflazione ha cominciato a crescere, dopo anni di livelli costanti; il il rischio è quello che all'inflazione si aggiunga anche la stagnazione, che è la peggiore delle condizioni economiche.

prevede lo scorrimento delle graduatorie degli allievi agenti di Polizia. Da molte parti c'è la richiesta di aumentare il numero e la presenza delle Forze di polizia, per la sicurezza delle città, per l'emergenza Covid, per l'ingresso dei profughi ucraini e per mille altre cose; evidentemente poi bisogna anche assumerle queste persone. Va anche bene l'approvazione di diversi emendamenti che riguardano il settore turistico. Ricordiamo che il turismo rappresenta il nostro petrolio,

riservato ai *tour operator* e alle agenzie di viaggio. E ancora la rottamazione-*ter*: questo è uno degli argomenti sui quali la Lega ha sempre insistito, perché, in assenza di un intervento, ciò avrebbe causato il *default* di tantissimi artigiani e commercianti (si parla di 600.000 persone). Quindi è una cosa assolutamente positiva. C'è stata anche la proroga dei termini per l'approvazione del rendiconto e del bilancio consolidato 2021 in materia di rendicontazione del Servizio sanitario regionale (un aiuto alle Regioni). C'è stato poi, durante la trattazione, un episodio che riguarda i contratti di somministrazione.

da tutta la Commissione, ad eccezione del Gruppo della Lega, che ha votato in modo contrario. Pensiamo infatti che in questo momento di grande crisi del lavoro occorra difendere il lavoro e non facilitare licenziamenti. *(Applausi)*. Ricordo che sono a rischio 110.000 posti di lavoro recentemente sono stati licenziati 450 interinali da Poste Italiane. Questo è quello che purtroppo è successo ed è incomprensibile, ma voglio ancora ricordare brevemente quello che non è stato fatto, c'era un emendamento del collega Arrigoni circa la qualificazione delle imprese, un emendamento non oneroso e importantissimo che ci hanno chiesto tutte le categorie del settore edile, perché avrebbe permesso di escludere tutte quelle imprese che sono nate come funghi senza personale, quella zona grigia nella quale poteva risiedere anche

perché avrebbe premiato gli imprenditori seri che con fatica continuano a stare in piedi e a dare lavoro per davvero. Vi erano poi altri emendamenti, come quello del collega Briziarielli, che prevedeva misure per gli organi preposti all'attività di vigilanza e controllo ambientale, o quello della senatrice Cantù sull'attività libero professionale del personale sanitario. possibile che con il lavoro così importante che è stato fatto, nonostante tutti i limiti di tempo, dettati della fretta o dalla situazione - come dicevo prima - anacronistica, non si riesca non si riesca a portare a termine l'*iter* di alcune proposte assolutamente buone e positive, perché non arrivano fisicamente, all'ultimo secondo, gli emendamenti. Su questa cosa dovremo intervenire

rappresentanti del Governo, colleghe senatrici e colleghi senatori, il mio intervento di oggi verterà su due punti: la soddisfazione per il passaggio di un emendamento che ritengo importante per aiutare i Comuni e la delusione per come sono andati i lavori emendativi del presente decreto-legge. Certo, ci sono tante cose positive nel decreto, altre che avremmo voluto correggere, altre che abbiamo corretto e altre che abbiamo introdotto, ma su una cosa possiamo essere tutti d'accordo questo decreto è ormai superato dalle situazioni in corso, la guerra in Ucraina, e dalle complessità acuite dal conflitto - acuite perché c'erano già prima - che impattano sugli italiani. Una fra tutte è il caro bollette, che è affrontato ma non è risolto in questo decreto e avrà bisogno di ulteriori interventi che sono stati peraltro già annunciati. L'intervento di questo decreto, con cui si stanziano 1,7 miliardi per il caro bollette, segue gli ulteriori 3,8 miliardi stanziati in legge di bilancio, ma sappiamo che servirà solo a tamponare la situazione esistente e che bisognerà intervenire in maniera strutturale e definitiva per risolvere il problema della dipendenza energetica dell'Italia dagli approvvigionamenti esteri. Proprio questa mattina il ministro Cingolani è venuto a riferire qui in Aula sulle problematiche relative al costo degli approvvigionamenti e sappiamo che dovremo agire sia sul fronte dell'aumento della produzione di gas italiano e dell'approvvigionamento da altri Paesi, sia sulla spinta per le rinnovabili, semplificando le procedure di installazione degli impianti. Cominciamo dalle parti positive: con un emendamento del MoVimento 5 Stelle da me presentato abbiamo dato una mano a una parte di quei 3.000 piccoli Comuni, su quasi 8.000, che subiscono da anni la mancanza di segretari comunali. Non ce ne sono a sufficienza, alcuni devono addirittura saltare da una sede all'altra, su quattro sedi. Ora non voglio entrare nel tecnicismo dell'emendamento, ma di fatto con la modifica da noi proposta i segretari di fascia C, quelli che sono abilitati ad esercitare nei Comuni fino a 3.000 abitanti, che sono - ricordo - il 56 per cento dei Comuni italiani, potranno esercitare anche nei Comuni fino a 5.000 abitanti, cioè il 70 per cento dei Comuni. Questo permette anche ai segretari già in servizio di aggregare più Comuni fino a tali limiti. Con questo emendamento, quindi, da subito più di 500 Comuni italiani potranno dotarsi finalmente di un segretario comunale, una figura cardine che assicura la direzione apicale degli uffici nel rispetto della legalità, una figura indispensabile per aiutare questi enti in un momento in cui il PNRR dovrà essere portato avanti. Questo è un primo passo, ma una soluzione definitiva andrà trovata. Come dicevo prima, il decreto porta all'interno un grande punto positivo del MoVimento 5 Stelle, anche se non posso definirla una vittoria, perché siamo amareggiati per quello che vedremo in seguito essere l'altra faccia della medaglia. Nel decreto il Governo ha inserito un emendamento che nasce dalla pressione esercitata nel mese scorso, soprattutto dal MoVimento 5 Stelle, immediatamente dopo la pubblicazione del decreto sostegni-*ter*. Nel provvedimento era stato introdotto il famigerato articolo 28, quello che di fatto bloccava tutte le cessioni successive alla prima dei crediti d'imposta dei *bonus* edilizi, fra cui quelli del superbonus. Il mercato si è immediatamente bloccato. Poste e tutti gli operatori bancari non hanno più rilevato i crediti questo stop è stato dato dal Governo sulla base della valutazione errata che la maggior parte delle frodi, quantificate in circa 4 miliardi, fossero imputabili al superbonus.

i 130 milioni sul totale di oltre 13 miliardi di euro di crediti d'imposta già richiesti stiamo parlando dell'1 per cento, una percentuale che potrei definire fisiologica, su cui certo bisogna intervenire, ma non bloccando, perché a questo punto con lo stesso criterio dovremmo smettere di far viaggiare gli autobus pubblici perché c'è qualcuno che non paga il biglietto. quindi, il Governo ha dovuto riconoscere di aver fatto un errore clamoroso, lo ripeto, clamoroso, perché ha preso una decisione che ha di fatto bloccato tutto - e lo si sapeva senza guardare ai dati specifici dei singoli *bonus*. Pertanto in fretta e furia, in base alle pressioni che ha ricevuto, ha dovuto emanare questo decreto trasposto in emendamento nel decreto sostegni-*ter*, che ha ripristinato le cessioni, anche se in maniera limitata. Ma il Governo, ed è questa l'altra faccia della medaglia, quella per cui sono e siamo delusi, non ha valutato - e poco importa se non ha voluto valutare o se non è riuscito a valutare - nessuno dei quasi 50 subemendamenti al decreto, emendamenti presentati da tutti i Gruppi politici, alcuni dei quali addirittura non onerosi, che avrebbero fluidificato il sistema. È chiaro che siamo in un periodo che possiamo definire di ingorgo normativo. Sappiamo che a breve sarà discussa una serie di provvedimenti fra Senato e Camera e come MoVimento 5 Stelle intendiamo riproporre le nostre soluzioni: continueremo a discuterle e a sottoporle al Governo e ai Ministeri. Dico chiaramente che a noi andrebbe anche bene se il Governo le valutasse, le facesse proprie e le inserisse direttamente nei provvedimenti, perché sono proposte che servono a facilitare la vita dei cittadini e delle imprese. proposto, per esempio, una soluzione per evitare il limbo in cui finiscono i crediti d'imposta che non vengono accettati dai soggetti cessionari. Avevamo proposto in particolare che, decorsi trenta giorni, in maniera automatica venissero rilasciati, così che il cedente potesse decidere per un'altra strada, magari anche per utilizzarli in compensazione fiscale, ma neanche un emendamento di buon senso come questo e a costo zero è stato valutato. valutato quello che avrebbe permesso agli istituti di credito di effettuare un'ultima e definitiva cessione nei confronti dei propri clienti per l'utilizzo nel pagamento dei propri debiti fiscali. Questo avrebbe permesso alle banche, specialmente alle piccole, che magari non comprano più perché sono vicine alla loro capacità fiscale, di evitare di essere sottoposte alle pressioni nelle riduzioni dei prezzi di acquisto dalle grandi banche, come credo che stia già accadendo. In quest'ultimo anno di legislatura andremo avanti praticamente solo per quella che un tempo era definita decretazione di urgenza e che ora possiamo definire decretazione normale nel senso statistico del termine. Se però non si trova un meccanismo per permettere al Parlamento di intervenire in maniera costruttiva, chi continuerà a farne le spese saranno i cittadini e le imprese. Qualsiasi azione da parte del Governo che, di fatto, riduca il dibattito parlamentare e l'analisi delle proposte emendative

Non sto qui a riproporle, ma mi auguro davvero che il Governo possa partire da questo documento per fare proprie le azioni che stanno a cuore *in primis* a cittadini e imprese e a praticamente tutto l'arco parlamentare, perché in tempi difficili occorre mettere da parte le aspirazioni personali e sintetizzarle in azioni che servono a far riprendere questo Paese e a farlo correre. Riuscire a portare a termine i progetti del PNRR è una sfida troppo importante che non possiamo perdere e l'apporto e la centralità del Parlamento, come ha anche ricordato il presidente Mattarella nel suo discorso di insediamento, è fondamentale.

che abbiamo presentato al Governo nello scorso febbraio su una circostanza rilevante come i decessi da Covid. Si tratta di un argomento sul quale si sarebbe dovuta impegnare una Commissione d'inchiesta, se ce l'avessero lasciata perché tutti i Parlamenti europei hanno messo a disposizione dei propri cittadini delle Commissioni di inchiesta parlamentare che facessero luce sui tanti aspetti della pandemia e dell'emergenza che ne è conseguita, ma non Ci sono le Regioni che in Italia hanno istituito Commissioni di inchiesta, ma il Parlamento no, perché c'è l'emergenza (questa è la motivazione per cui non si può istituire una Commissione d'inchiesta parlamentare). Ebbene, i cittadini giudicheranno al riguardo. Uno dei primi temi che una ipotetica Commissione d'inchiesta avrebbe dovuto affrontare è l'eccesso di mortalità nel nostro Paese rispetto al panorama europeo: i nostri morti per Covid sono i più numerosi.

mazzata all'economia nazionale, perché il nostro PIL è quello che ha subito la maggiore decurtazione. Su questi due dati, Presidente, abbiamo interrogato il ministro Speranza e vorremmo avere risposta, posto che proprio su «la Repubblica» che cita un rapporto di «The Lancet», che rispetto ai temi sanitari è una sorta di Vangelo, basato su uno studio mondiale che analizza puntualmente i decessi per Covid di tutto il mondo e rileva che in Italia, rispetto a quelli registrati che sono oltre 160.000, ce ne sarebbero 120.000 in più.

Presidente, colleghi, nei giorni scorsi ho presentato - all'attenzione del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - un'interrogazione al fine di chiedere chiarimenti ed eventuali e conseguenti urgenti interventi in autotutela con riferimento alla decisione di non ritenere ammissibili due richieste di finanziamento formulate nell'interesse delle aree interne della Campania e in particolare per il distretto idrico Calore Irpino ovvero per le province di Benevento e di Avellino, per un importo pari a circa 56 milioni di euro, con riguardo all'avviso pubblico avente ad oggetto la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresi la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti. Tenuto conto che, per esperienza personale - come magari avrà anche sentito dire - le interrogazioni non hanno quasi mai risposta, ho ritenuto di far giungere la mia voce forte e chiara al Ministro attraverso questo intervento di fine seduta. Calore Irpino rappresenta, con le sorgenti di Caposele, Cassano Irpino, Cesinali, Serino ed altre, presenti nella provincia di Avellino, e con la Diga di Campolattaro presente nella provincia di Benevento, uno dei bacini idrici più importanti d'Italia e d'Europa dai quali proviene la risorsa idrica servita oggi e che verrà servita in misura sempre maggiore in futuro a milioni di cittadini tra Puglia e Campania. Tale area interna della Campania non può essere solo depredata della propria preziosa risorsa idrica senza ricevere quantomeno la possibilità di migliorare l'efficienza delle reti di distribuzione dell'acqua a servizio del territorio. Non si può condividere pertanto che tutto venga risolto con la laconica motivazione che la proposta non risulta ammissibile, atteso che l'EGA ha dichiarato di non aver ancora ultimato le verifiche in ordine alla conformità dell'affidamento. L'ente idrico campano aveva fornito anche riscontri, rassicurazioni e proposte al Ministero e in ogni caso è assurdo che, pur in presenza di proposte progettuali di ottimo livello, non si ritenga neanche di valutare le stesse nel merito

prescindere da un prossimo eventuale cambio di gestore che potrebbe concretizzarsi a seguito di gara e nel subentro di un nuovo soggetto ai due proponenti Alto Calore e Gesesa. Al Ministro dico che i finanziamenti sono per il bene dei cittadini e del territorio e non delle società che hanno redatto i progetti, ed è a quei cittadini e a quei territori che il Ministero farebbe un gravissimo danno. Chiedo che Chiedo quindi che sia effettuata una valutazione nel merito delle due proposte progettuali in questione con la relativa attribuzione di punteggio e l'inserimento nella graduatoria. Poi, si vedrà se le proposte si riveleranno degne di ricevere l'intero finanziamento

«Sono la mamma di una ragazza di quindici anni, N , una ragazza sportiva, sana che fino al 2 di settembre 2021 aveva un sogno, fare la ballerina. Per questo frequentava lontano da casa un'accademia di danza per la quale però sarebbe servito il *green pass* per poter continuare a studiare. Decide dunque di fare la prima dose di Moderna, quella mattina è iniziato il nostro incubo. Pochi minuti dopo l'inoculazione, N inizia a star male: mal di testa, male al braccio e una debolezza che si propagava col passare dei minuti. Viene stesa su un lettino e portata al pronto soccorso. Man mano che passavano le ore, N non si reggeva nemmeno più in piedi. Due visite neurologiche, analisi e TAC rivelano niente di anormale e quindi viene sottoposta a visita neuropsichiatrica. La mattina dopo viene dimessa in uno stato ancora pietoso, con la diagnosi di ansia. La porto a casa in braccio e per due settimane ho dovuto imboccarla e aiutarla in tutto, perché lei non riusciva a muoversi. Il braccio non si alzava più e le gambe non reggevano. I medici mi rassicuravano che sarebbe passato presto e di darle paracetamolo. Prenoto una visita neurologica, dove mi viene consigliato il ricovero. Una settimana in ospedale, con flebo di paracetamolo e diverse visite psichiatriche senza alcun miglioramento. Chiedo che le venga somministrato cortisone, almeno per far passare il dolore al braccio e vedere se si muove. Niente, mi viene negato tutto. Per loro la diagnosi è chiara: deve andare dallo psichiatra. Ma io conosco bene mia figlia. Non è pazza e se dice di star male sta male davvero. La faccio dimettere e la porto a casa, senza alcun miglioramento. In quel momento mi sono ritrovata davanti a un buco nero: chi mi aiuta? A chi mi rivolgo? Siamo ormai a novembre e N ha già perso mesi di scuola di danza. Decido di andare al centro vaccinale a chiedere aiuto. Fortunatamente, lì ho trovato medici che hanno capito la situazione, confermandomi che mia figlia stava male davvero, ma che purtroppo non sapevano cosa fare. Si sono susseguite varie visite neurologiche, allergologiche e cardiologiche. Il risultato è che N ha un disturbo funzionale neurologico, causato dal vaccino, e probabilmente ha avuto anche la miocardite. Dovrà fare ancora risonanza magnetica per conferma*.

Presidente, colleghi presenti in Aula, io sono qui a ricordare che una delle responsabilità concrete del Governo è rispondere alle interrogazioni dei parlamentari. In questo momento, sono qui a ricordare con precisione due interrogazioni, che hanno come oggetto specifico la capacità e la possibilità di intervenire sul fumo,

per non rimanere fuori dalla concretezza della mia denuncia. Sono elementi che concorrono a creare una condizione

capaci di illuminare, prima, di più e meglio, questa patologia, che rappresenta comunque una delle maggiori cause di mortalità ancora oggi. Tra i fattori che che predispongono al cancro, sapevamo tutti che c'era il fumo, ma era escluso che il fumo potesse riguardare anche le nuove forme, i nuovi modelli di fumo. Ciò è tanto vero, signor Presidente, ed è il motivo per cui da tempo porto avanti questa battaglia, che il fumo da tabacco riscaldato gode di un'agevolazione fiscale, che raggiunge il 70 per cento, con la premessa che questo fumo non nuoce alla salute. Il documento di ieri del Parlamento europeo, documento approfondito, analitico, concreto e preciso mostra che questa relazione esiste.

Signor Presidente, l'ultima volta che ho trattato questo tema ho detto che speravo di non doverlo più fare; ho lasciato correre parecchi incidenti, ma oggi sono costretto a riprendere un tema

Era la seconda volta: circa un anno prima aveva demolito la macchina, ma se l'era cavata, in questo parco del Gargano dove forse manca una corretta gestione faunistica (essendo un parco) e succedono cose di questo genere, come in tante altre parti d'Italia. d'Italia. Desidero ricordarlo insieme a tutti gli altri. Non c'è più, è morto. Un paio di cinghiali si sono fatti male. Qualche sera fa un nostro collega, il senatore Briziarelli, ha rischiato di fare la stessa fine; ne è venuto fuori per miracolo, un cinghiale si è fatto male. Noi stiamo dalla parte di Gino Turco, imprenditore morto che non c'è più, e dalla parte del senatore Briziarelli. Non stiamo dalla parte dei cinghiali.

che venga affrontato anche il problema della presenza degli animali e dei cinghiali all'interno dei grandi centri urbani. Siamo andati al voto su questo tema e la compagine politica di cui ho parlato prima ha bocciato questa proposta. Lo dico da genovese,

Grazie Signor Presidente, onorevoli colleghi, alla crisi legata alla pandemia, già di per sé estremamente gravosa, si è aggiunta la crisi russo-ucraina che ci sta facendo ripiombare in un contesto di paura e instabilità. condizione deriva non solo da effetti strettamente connessi al conflitto e alle sofferenze causate al popolo ucraino, a cui va il nostro accorato pensiero, ma anche dai risvolti economici e sociali. Mi riferisco al rincaro dei prezzi delle materie prime e dei combustibili, che tutti viviamo sulla nostra pelle. del 10 marzo 2022 la quotazione record per gasolio e benzina in Italia, salita a 2,5 euro al litro, con il prezzo del diesel arrivato a superare quello della benzina. Se da un lato questo innalzamento dei prezzi è collegato al conflitto in atto, da un altro è frutto di una psicologia perversa che si impernia sulla paura e sulla speculazione. Proteste e scioperi si stanno quindi moltiplicando giorno per giorno in tutto il Paese, aggiungendo disagi ai disagi. In Italia l'80 per cento della merce viaggia su gomma e con il costo dei carburanti a questi livelli la distribuzione rischia di bloccarsi. Massima solidarietà agli autotrasportatori che denunciano a gran voce insostenibili perdite. oltre 2.000 euro mensili, che riguardano non solo i vari rincari, ma anche altri oneri che da anni attendono correttivi risolutivi, restando però puntualmente inevasi. Stessa sorte per i pescatori, fermi in porto da giorni perché non ritengono conveniente uscire in mare per pescare in quanto avrebbero spese doppie e sanno di non potersi poi rifare sul consumatore finale. Come dargli torto. per gli agricoltori che lamentano l'aumento repentino dei prezzi di materie prime indispensabili per l'attività, oltre che del carburante. Materie prime quali sementi e concimi, per non parlare dei mangimi per il settore zootecnico. Questa situazione si va a sommare alla diminuzione della disponibilità di cereali da Paesi quali Canada e Ungheria, da cui importiamo materia prima indispensabile all'industria molitoria italiana, che non sarà più in grado di garantire la produzione nei volumi richiesti dal mercato. La drammaticità di questo scenario sta esacerbando una situazione già critica e si paventa il rischio di ritrovarci in un vero e proprio *tsunami* su scala europea, le cui conseguenze nefaste arriverebbero a cascata su molti settori e non solo nelle filiere direttamente collegate. È urgente e necessario intervenire congiuntamente a livello europeo per intavolare una discussione sul *recovery* emergenziale, al fine di garantire celermente misure e interventi per assicurare stabilità e prevenire situazioni di crisi. indispensabile porre regole chiare sul costo delle risorse energetiche per eliminare pericolose derive capaci di mettere in di mettere in ginocchio il tessuto produttivo destabilizzando pericolosamente l'intero assetto economico, come da tempo ripetono a gran voce tutti gli operatori del settore. Come MoVimento 5 Stelle siamo pronti a fare tutto il possibile per dare il massimo supporto alle categorie in difficoltà.

ed approvato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022 n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, di salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi